è una grande occasione non solo per ricordare lo statista che, con il suo impegno e con le sue intuizioni, è stato uno degli artefici dell'Unità, ma anche per un'ulteriore riflessione sugli eventi fondativi dello Stato nazionale. Pur «lontano dalla tradizione culturale italiana», secondo la definizione di Federico Chabod, e più attento alle grandi trasformazioni che investivano l'Europa occidentale, nel corso degli anni Cavour maturò una grande attenzione nei confronti della Penisola, i cui destini vedeva legati a quelli continentali: e il piemontese che si sentiva europeo grazie alla formazione cosmopolita divenne presto italiano, come ha ricordato Rosario Romeo. Mosso da una fede quasi religiosa nel progresso dell'umanità, riteneva che la libertà politica e quella economica, intimamente legate ai suoi occhi, dovessero essere il motore dell'opera di «incivilimento» delle società. La libertà di commercio e lo sviluppo delle banche e delle ferrovie, a suo avviso, avrebbero generato una prosperità diffusa e aperto all'Italia le porte del mondo moderno, ponendo fine all'inquietudine che tormentava il Paese. L'unificazione economica e il tramonto dell'egemonia asburgica erano quindi indispensabili alla formazione di uno Stato nazionale, a sua volta premessa necessaria al consolidamento di una società liberale. Lasciando agli storici il compito di individuare l'ampiezza del disegno politico originario di Cavour - se cioè avesse in mente fin dai primi atti di governo una vera e propria «idea italiana» e dunque un progetto politico esteso all'intera Penisola è certo comunque che egli, pur ritenendo «essere la storia una grande improvvisatrice», come affermò in un discorso parlamentare del 1857, non si fece sorprendere dagli avvenimenti. Convinto della necessità di attuare profonde riforme per evitare dannose rivoluzioni, avviò nel Regno di Sardegna un rinnovamento dei gangli vitali dello Stato, anche mediante un massiccio avvicendamento del personale, soprattutto di vertice. In questo modo favorì la creazione dei quadri politici e amministrativi della nuova Italia, pur ancora di là da venire, mentre le innovazioni economiche e finanziarie, non disgiunte da un utilizzo ardito del debito pubblico, aprirono la strada alla formazione di un ceto dirigente e di una realtà imprenditoriale che assicurarono il consenso sociale all'accordo politico del «connubio», da lui considerato il più bell'atto della sua vita politica. Nell'operazione di rimodellamento dello Stato e di ricerca del consenso sociale, fu attento a ricercare e ottenere l'appoggio della nuova realtà dell'opinione pubblica, alla quale spesso si richiamava, come a «una specie di fumo» che «tosto o tardi trasformandosi in vapore solleva i maggiori ostacoli e vince le maggiori difficoltà». Consensi minori raccolse invece presso la popolazione la sua politica in materia ecclesiastica e soprattutto la soppressione degli ordini contemplativi e mendicanti e l'incameramento dei loro beni, giustificati - nel discorso parlamentare del 17 febbraio 1855 - sia da considerazioni di natura finanziaria sia dalla convinzione di saper discernere quali fossero gli ordini religiosi ancora «utili» alla Chiesa e alla società. I grandi mutamenti sullo scenario internazionale gli consentirono di uscire dall'*impasse* della politica interna, nella corretta convinzione di poter ottenere risultati concreti solo agendo sul piano europeo, dove stava mutando il rapporto di forze fra rivoluzione e conservazione. Abile nel giocare su più tavoli nei momenti decisivi - il Congresso di Parigi, l'armistizio di Villafranca, la spedizione dei Mille e l'occupazione delle Marche e dell'Umbria pontificie - ebbe la felice intuizione di perseguire una «rivoluzione italiana con un re» tanto temuta invece dal repubblicano Giuseppe Mazzini - per superare gli assetti territoriali fissati al Congresso di Vienna ed evitare al contempo il rischio di una deriva sovversiva. In questo modo riuscì a «costituzionalizzare» la rivoluzione, anche assumendo rischi che non escludevano l'azzardo di fronte a fattori non previsti, ma avendo sempre come stella polare il Parlamento. «Io credo che con il Parlamento si possano fare molte cose che sarebbero impossibili per un potere assoluto», scrisse nell'ottobre del 1860; un'affermazione che tuttavia non escludeva comportamenti più audaci, come in occasione degli accordi di Plombières, quando confidò al fidato collaboratore Costantino Nigra: «Controfirmando un trattato segreto che comporta la cessione di due province, io commetto un atto altamente incostituzionale», aggiungendo tuttavia: «Credo di poter garantire moralmente l'adesione del Parlamento. Il re e io non ne dubitiamo». L'annessione del Mezzogiorno fu poi il suo capolavoro politico. Duttile e pragmatico, di fronte a vicende il cui esito non era affatto scontato, riuscì a tenere sotto controllo tutte le forze in campo, eterogenee e fra loro divergenti, e a indirizzare gli avvenimenti verso la conclusione unitaria, così imprevista da fargli dichiarare, nel dicembre 1860: «Ora che la fusione delle varie parti della Penisola è compiuta, mi lascerei ammazzare dieci volte prima di consentire a che si sciogliesse». Si accinse quindi ad affrontare le grandi questioni sorte con l'Unità, di cui vedeva la complessità: «Il mio compito» - ebbe a scrivere nel febbraio 1861 - «è più laborioso e penoso ora che per il passato. Costituire l'Italia, fondere insieme gli elementi diversi di cui si compone, mettere in armonia il nord e il mezzogiorno presenta tante difficoltà quanto una guerra contro l'Austria o la lotta per Roma». Più che di fare gli italiani, che esistevano da secoli come nazione, si trattava di fare l'Italia, cioè di costruire lo Stato unitario nelle sue articolazioni. Potenzialmente favorevole a forme di autogoverno delle autonomie locali, non intendeva mettere a repentaglio l'Unità faticosamente conseguita e, a scanso di equivoci, dichiarò in Parlamento: «Dopo tutto quello che d'impensato e d'insperato avvenne nella penisola, ognuno indovina che noi non siamo federalisti». Si arenò dunque l'idea di una «scentralizzazione» e il modello dello Stato burocratico e centralizzatore prevalse per ragioni politiche, legate soprattutto alla grande resistenza all'annessione in atto nell'ex Regno delle Due Sicilie. Cavour, infatti, era molto scettico sull'opportunità di salvaguardare l'autonomia dell'antico regno, come si espresse in una lettera scritta al fedele collaboratore Costantino Nigra due settimane prima della proclamazione del Regno d'Italia, dove giudicava necessaria «la distruzione di quella fatale autonomia» del Mezzogiorno «che rovinerà l'Italia se non ci rimediamo». Convinto, come tanti, della ricchezza naturale delle regioni meridionali, a suo giudizio abbrutite da secoli di malgoverno, confidava negli effetti positivi che sarebbero derivati dall'unificazione del mercato nazionale, ma non poté assistere alla disillusione degli anni postunitari e alla nascita della Questione meridionale. Quanto alla Questione romana, capitolo della più ampia questione cattolica, nei discorsi parlamentari del marzo 1861, dopo aver sostenuto che solo Roma - dove però non volle mai recarsi - poteva essere la capitale del nuovo Stato unitario perché era l'unica città che non avesse memorie solo municipali, proclamò la formula «libera Chiesa in libero Stato», cui era sottesa la scelta della separazione. Questa impostazione, com'è noto, è stata superata nel tempo da una politica di conciliazione che ha prodotto fra le due istituzioni rapporti equilibrati e fondati sulla collaborazione e sul rispetto. Cavour scomparve il 6 giugno 1861, all'età di cinquant'anni, senza poter contribuire allo sviluppo e al consolidamento di quella costruzione politica, non esente da crepe ma tuttora salda, che in modo determinante ha contribuito ad erigere. Alla sua memoria, l'Aula del Senato rende oggi omaggio, per la testimonianza di un uomo delle Istituzioni, di autentico e coraggioso servitore dello Stato, che ha accettato di lavorare per l'Italia, sapendo che altri avrebbero raccolto i frutti della sua instancabile e prestigiosa opera.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricordiamo il conte di Cavour a 150 anni dalla morte. Il 17 marzo scorso abbiamo celebrato i 150 anni dell'Unità d'Italia. Due date sulle quali è scolpita la nostra storia nazionale, massimamente tributaria a questo colosso della politica di cui, mi si conceda il passaggio, come parlamentare piemontese posso dirmi particolarmente fiero. Ma Cavour non è solo un monumento dei piemontesi: è stato il vero artefice della Nazione e non è un caso che ad averne scritto una fondamentale biografia sia stato l'avellinese Italo De Feo. Ora, i 150 anni dell'Unità ci hanno fatto un ulteriore regalo: la ristampa di questa preziosa biografia recentemente presentata a Palazzo Giustiniani, presente la figlia, senatrice Diana De Feo, e gli illustri colleghi Gaetano Quagliariello e Luigi Compagna. Non potendo, per più di un motivo, ripercorrere qui la vicenda storica e politica del conte Cavour, mi limiterò a disegnare i tratti essenziali che definiscono, un secolo e mezzo dopo la sua scomparsa, le qualità dello statista. È un uomo profondamente moderno che piacerebbe a tutti coloro che oggi e negli anni passati hanno propugnato la politica del fare. Come uomo di governo interpretò al meglio questo concetto del fare, soprattutto con i grandi investimenti industriali e infrastrutturali dalle ferrovie, alle grandi vie di comunicazione, comprese quelle con i Paesi transalpini; in particolare mi piace qui ricordare oggi, per ovvie ragioni di attualità, la realizzazione del traforo ferroviario del Frejus e del Colle di Tenda. Uomo straordinariamente moderno, quindi, introdusse la forma del partenariato pubblico e privato per la realizzazione delle infrastrutture, in particolare le opere ferroviarie. Uomo pragmatico, riuscì a conciliare e ad interpretare al meglio quello che oggi tutti vorrebbero che si realizzasse: innovazione e ricerca. Ma egli la fece attraverso le iniziative concrete di industrializzazione del nostro sistema economico, ma anche nel rivoluzionario e produttivo modo di affrontare i temi dell'agricoltura, introducendo nuove coltivazioni, facendo opere di bonifica e costruzioni di canali di irrigazione. Per Cavour un'agricoltura ricca e moderna era alla base per lo sviluppo dell'industria. Favorì la creazione di un'industria siderurgica e il potenziamento di quella tessile, impiantò in pratica dal nulla la rete telegrafica. Principalmente Cavour esaltava gli investimenti infrastrutturali come strumento di progresso civile al quale, piuttosto che alle sommosse, era affidata la causa nazionale. Egli a tale proposito mise in rilievo l'importanza che avrebbero avuto due linee ferroviarie: la Torino-Venezia e la Torino-Ancona. Il commercio venne favorito in ogni modo e la realizzazione di una vera marina mercantile fece rifiorire il porto di Genova. Camillo Benso aveva infatti fede nel progresso che era sopratutto intellettuale e morale, poiché risorsa della dignità e della capacità creativa dell'uomo. A tale convinzione si accompagnava l'altra, che la libertà economica è causa di interesse generale destinata a favore tutte le classi sociali. Il vero progresso di una Nazione non è da ricercarsi nel *welfare*, ossia nello Stato sociale, bensì nel dare lavoro e quindi dignità alle persone. Nel maggio del 1832, a ventidue anni divenne sindaco di Grinzane, carica che mantenne per 16 anni, fino al febbraio del 1849. Camillo Benso conte di Cavour è stato in grado di cogliere con incredibile tempestività tutte le occasioni offerte dalle vicende internazionali ad una potenza di secondo ordine come il Regno di Sardegna. Ha avuto l'abilità di tenere a bada un sovrano che, pur avendo confermato e difeso lo Statuto, aveva la tendenza istintiva a non limitarsi a regnare, ma a cercare con ogni mezzo di condizionare l'attività di governo. È stato in grado di cavalcare ed al tempo stesso incanalare nell'alveo delle regole del sistema costituzionale (allora niente affatto consuete) una forza della natura come quella rappresentata da Giuseppe Garibaldi. Ha marginalizzato le forze antisistema, rappresentate da un lato dal mondo clericale e reazionario, dall'altro dalla sinistra mazziniana, repubblicana, usando con sagacia solo le armi della politica e non quelle, più facili per l'epoca, di un autoritarismo di stampo illiberale. Cavour era un uomo che sapeva più e meglio di tanti altri come la politica fosse un'arte da realizzare con un pragmatismo e un realismo non condizionati da scrupoli di sorta ma sempre ancorata a grandi principi. per Camillo il principale di questi principi era quello della libertà, che era l'unica istanza di innovazione e di progresso dopo l'era dell'assolutismo restaurata ed imposta all'Europa ed all'Italia con il Congresso di Vienna, ma che, per non essere astratto, schematico e pretesto di illiberalità, come prima l'esperienza del biennio del Terrore della Rivoluzione francese e poi il dispotismo napoleonico avevano insegnato, doveva essere attentamente preservata da qualsiasi degenerazione. Per Cavour questo principio di libertà andava applicato ovunque: nell'economia, dove la battaglia liberale si doveva manifestare con una legislazione tesa a favorire il libero commercio eliminando dazi, norme protezioniste e qualunque ostacolo alla circolazione delle merci e delle idee, secondo gli insegnamenti del più classico liberismo di scuola anglosassone. Nei rapporti internazionali, in cui proprio in nome di uno spirito di libertà che non doveva essere solo degli individui ma anche degli Stati, il suo sforzo principale fu di ribaltare la tradizionale subordinazione degli Stati italiani, in particolare del Regno di Sardegna, alle grandi potenze europee e di rendere prima il Piemonte e successivamente lo Stato unitario in grado di conservare una libertà di movimento sul piano interno ed internazionale, tale da renderli capaci di sfruttare al meglio le incertezze e le debolezze degli Stati europei dominanti. Anche se nel marzo del 1860 - in realtà il Trattato fu postdatato giacché la firma avvenne nel gennaio 1859 1859 - con il Trattato di Torino sancì l'annessione della Contea di Nizza e della Savoia alla Francia. E questo per un cuneese in particolare è stato un contributo lacerante pur nobilitato dal suggello dell'Unità nazionale. Il conte di Cavour aveva la sua ferma volontà di considerarsi, anche con il Re, non un suddito ma un cittadino, consapevole dei diritti e della dignità conseguiti con il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Nei rapporti con la Santa Sede, secondo Cavour serve realismo, pragmatismo e capacità di mediazione. Ma serve soprattutto assoluta fedeltà ai valori di libertà. Quei valori che oggi come allora dovrebbero rappresentare la sola ed unica stella polare della politica nazionale. Si racconta che le ultime parole pronunciate da Cavour siano state «l'Italia è fatta, è salva!». E sulla base di queste ultime battute si sostiene che la vera eredità lasciata agli italiani dal conte sia stato il suo contributo determinante alla formazione dello Stato unitario. La considerazione è corretta. Ma il capolavoro politico di Cavour, quello che dovrebbe ispirare i dirigenti politici di oggi e che invece viene contestato e considerato come la matrice di quel trasformismo ritenuto vizio congenito e mortale delle classi politiche italiane, è il famoso «connubio» parlamentare tra i liberali moderati vicini al conte ed i liberali progressisti di Rattazzi, cioè la formazione di una maggioranza ampia di moderati di diversa gradazione in grado di dare stabilità ad un governo difendendolo dagli attacchi delle forze antisistema. Grazie a quell'invenzione cavourriana, la destra storica e, successivamente, il centrosinistra riuscirono in un capolavoro politico: a stemperare progressivamente la «Questione romana» ponendo fine all'autoemarginazione dei cattolici dalla vita pubblica del Paese; a disinnescare il potenziale esplosivo dei mazziniani e dei garibaldini trasformandoli nella stragrande maggioranza in strenui difensori dello Stato di diritto; a scongiurare il pericolo che l'Unità si compisse all'insegna della democrazia autoritaria. autoritaria. La domanda, a questo punto, è: che cosa il conte avrebbe potuto fare per l'Italia se nei suoi confronti la vita fosse stata meno avara di anni? Ci restano i suoi insegnamenti, una lezione che dobbiamo tenere viva in questa nostra Aula e nell'intero Parlamento. Cavour è stato definito «dittatore parlamentare». C'è del vero in questa affermazione, ma noi dobbiamo trarne il significato più alto. Lo statista era un uomo del fare, ma anche un uomo del dialogo e un maestro nel difficile esercizio della diplomazia e delle relazioni tra i gruppi che compongono un'assemblea elettiva. Discuteva, trattava, mediava e raggiungeva il risultato. Per lui, sopra tutto, contava l'interesse nazionale. Per questo sarà ricordato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, avere la pretesa di esaurire nel tempo di dieci minuti la complessa e articolata personalità di Cavour è un po' come immaginare l'alba di una giornata senza poter raccontare appieno quali e quanti eventi l'hanno potuta riempire. Eppure mi piace condividere qui, in quest'Aula, in quest'anno carico di significati storici, una riflessione ad alta voce attorno a ciò che è stato, cosa ha rappresentato e quale messaggio ci trasmette oggi l'uomo, il politico, lo statista Cavour. Cavour nasce il 10 agosto 1810 a Torino, secondogenito del marchese Michele e della ginevrina calvinista Adele di Sellon, da cui eredita valori come l'etica del lavoro e la libertà di coscienza.

grazie all'educazione familiare, spinto dal profondo e crescente convincimento che i progressi economici e la politica sono strettamente correlati, decide di viaggiare nei Paesi europei per studiare da vicino gli effetti della rivoluzione industriale in Gran Bretagna, Francia e Svizzera. A Parigi ha modo di frequentare le principali istituzioni pubbliche, i più importanti intellettuali dell'epoca e non sarà inutile. A Londra si interessa non solo alla vita politica e culturale, ma anche alle profonde innovazioni tecniche. di questioni sociali e sviluppa il sempre più crescente interesse per il libero scambio. Cavour riteneva che il valore della nazionalità risiedesse nel connubio tra libertà economica che è causa di interesse generale ed è destinata a favorire tutte le classi sociali - e il progresso intellettuale e morale, frutto della dignità e capacità creativa dell'uomo. Questa grande ammirazione per la società inglese e francese lo porta a studiare in modo approfondito Smith, Malthus, Guizot e Tocqueville, di cui poi avrebbe applicato i precetti trasformando il Piemonte in quello Stato moderno che solo tramite il respiro europeo da lui fornitogli, si sarebbe potuto presentare come centro di aggregazione delle future istanze nazionali italiane. Secondo lo statista, lo sviluppo dei lumi e il progresso civile, senza alcun bisogno di sommosse popolari, avrebbero creato una crisi politica di cui l'Italia doveva approfittare. Rientrato in Piemonte nel 1835, si interessa di economia e applica sul territorio le esperienze acquisite nei viaggi all'estero. La fondazione nel dicembre 1847 della testata liberale e moderata «Il Risorgimento» segna l'avvio del suo impegno politico e qui si prende carico di attuare una profonda ristrutturazione delle istituzioni piemontesi e di istituire nuove riforme liberali, che avrebbero permesso al Regno sabaudo di uscire dall'arretratezza economica e di intraprendere quella via di industrializzazione che i grandi d'Europa stavano già percorrendo da più di mezzo secolo. fu eletto deputato, entra nel Governo D'Azeglio come Ministro dell'agricoltura prima e delle finanze poi. Cavour provvede a rinnovare il sistema fiscale, a potenziare il sistema bancario e collabora all'istituzione di una banca nazionale. Il grande merito dello statista italiano credo fu quello di saper proporre una politica di riforme che contava sull'appoggio della classe dirigente piemontese: la borghesia. Infatti, privo di fiducia nell'aristocrazia nella quale trovava le sue origini, vedeva nella classe sociale capitalistica lo stesso universo aperto «che solleva i poveri ed abbassa i ricchi», che percepiva anche Guizot, ma che doveva farsi carico degli interessi della comunità ponendosi come mediatrice sociale. Non bisogna però confondere il riconoscimento della necessità di cambiamento di cui l'Italia aveva assoluto bisogno con l'adesione alle idee rivoluzionarie di Garibaldi né a quelle repubblicane di Mazzini, che non coincidevano in nulla con l'ideologia cavouriana iniziale. il Primo Ministro sabaudo si decise solamente durante la Seconda guerra d'indipendenza ad accettare quell'unità d'Italia tanto agognata da Mazzini. Cavour, piemontese anzitutto, mirò ad ingrandire il Piemonte per le vie tracciate dall'esperienza del 1848 assecondando l'ambizione di Carlo Alberto, ma quando si accorse che si doveva e si poteva ottenere di più non esitò a farsi italiano e a mettersi risolutamente alla testa del movimento unitario. unitario. Mi interessa sottolineare questi dati: ingrandire il Piemonte (tesi di Cavour), fare l'Italia (ideale di Mazzini). E fu sempre grazie a questa capacità di rielaborazione degli estremi che fu nominato nel 1852 Capo del Governo, in seguito a quella manovra politica, ironicamente definita dai suoi avversari «connubio», siglando un accordo con Rattazzi allo scopo di formare un nuovo Governo capace di mirare alla realizzazione di riforme che escludessero le ali estreme del Parlamento. Nasce così il centrismo che fa del centro quel luogo politico, che spostandosi un po' a destra o un po' a sinistra in base alle esigenze, governerà il Piemonte e poi dal 1861 fino all'ultimo decennio del XX secolo il neo costituito Regno di Italia. Cavour, dopo aver rafforzato su tutta la linea il Regno sabaudo, si dedicò ad un'audace, spregiudicata politica estera che aveva come obiettivo quello di far uscire il Piemonte dall'isolamento in cui versava, esprimendo finalmente i suoi ambiziosi Il primo passo da fare era quello di imporre il problema italiano all'attenzione europea e a ciò Cavour mira con tutto il suo ingegno. Fu per questi motivi che fece partecipare il Piemonte alla guerra di Crimea e che cercò l'alleanza con la Francia di Napoleone III nel 1858, che si impegna a sostenere militarmente il Piemonte qualora sia attaccato da potenze straniere. Poco dopo (nel 1859), a causa di reiterate provocazioni piemontesi ai confini con la Lombardia austriaca, l'Austria dichiara guerra all'Italia. Scoppia così la Seconda guerra di indipendenza, che annette al Piemonte non solo la Lombardia ma anche l'Emilia e la Toscana, che nel frattempo si sono ribellate ai loro governi e hanno votato l'annessione allo Stato sabaudo. In questo periodo Cavour apre le trattative con Garibaldi che era stato, insieme a Mazzini, uno dei protagonisti della Repubblica romana del 1849, il quale nonostante sia di fede repubblicana accetta di collaborare con Cavour pur di raggiungere l'obiettivo dell'unificazione d'Italia. È il tempo della spedizione dei Mille. Garibaldi in pochi mesi arriva dalla Sicilia a Napoli e tenta di proseguire verso Roma, ma Napoleone III fa sapere che se si tocca Roma lui dichiarerà guerra ai Savoia. Vittorio Emanuele quindi, su indicazioni di Cavour, scende col suo esercito verso Sud per fermare Garibaldi. Non passa sul Lazio ma sull'Abruzzo e le Marche che, insieme all'Umbria, subito chiedono l'annessione. È il 1861, è l'unità d'Italia. Si realizza il sogno risorgimentale, l'apoteosi dell'abilità diplomatica di Cavour si fonde con l'eroismo dei Mille, delle Cinque giornate di Milano, delle Dieci giornate di Brescia. Termina la lunga giornata di Cavour, vissuta intensamente, dall'alba al tramonto, senza tregua, senza soste, sempre sulle barricate delle cose difficili: giusto il tempo per cogliere il frutto di una fatica, e la storia lo porta con sé! Quanti interrogativi, quante riflessioni, quanti messaggi! Lascio all'Aula e a chi ascolta un tratto del suo agire, un impegno mantenuto, quasi un monito, citando le sue parole: «Dovessi rinunziare a tutti i miei amici di infanzia, dovessi vedere i miei conoscenti più intimi trasformarsi in nemici accaniti, non fallirei al dover mio, non abbandonerei mai i principi di libertà ai quali ho votato me medesimo, del cui sviluppo ho fatto il mio compito, ed a cui per tutta la mia vita sono stato fedele». E vi pare poco?

Presidente, la ringrazio e ringrazio anche per questa seduta, perché penso che la commemorazione del Cavour sia il giusto complemento alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia; non solo perché Cavour è stato di gran lunga il maggior artefice dell'Unità e nemmeno solo perché il conte aveva un profilo biografico di interesse tale che ha negli anni suscitato l'attenzione degli storici stranieri ancor più che degli storici italiani. A questo proposito vorrei leggere solamente poche parole dell'*incipit* di una delle più belle biografie, scritta da Italo De Feo, il padre della nostra collega realtà, ancor più che una biografia è un vero e proprio romanzo, soprattutto sulla formazione del conte: «Ebbe molte esperienze: fu beniamino di graziose fanciulle e donne, affarista e giocatore d'azzardo, gentiluomo di campagna e maestro di agricoltura, esperto di economia e finanza, studioso di storia e di problemi sociali. Amò la tavola e la musica, si distinse nelle discipline matematiche, fu buon oratore e infine giornalista e scrittore efficace». Sono poche frasi, che magari oggi oggi susciterebbero l'attenzione perversa di qualche procuratore, ma che invece racchiudono il profilo di un uomo eccezionale sotto tutti gli aspetti. la vicenda di Cavour, al di là della sua biografia, abbia un nesso profondo con questi 150 anni della nostra storia, perché si interseca con la difficoltà del fare l'Italia e del fare gli italiani. Vedete, signor Presidente e colleghi senatori, in realtà noi celebriamo oggi una storia che è stata una storia difficile e molto spesso anche una storia drammatica. L'unità italiana può considerarsi a tutti gli effetti un miracolo della politica e ci fa comprendere come la politica, oltre che una brutta cosa, come oggi viene spesso - troppo spesso - rappresentata,

C'erano difficoltà internazionali che, al di là del genio del conte in questo ambito, non possono essere rappresentate come spesso ha colpevolmente Non c'era nemmeno l'accordo della Francia, che pensava piuttosto ad un'unità che riguardasse solamente il Nord,

Esistevano difficoltà note nel fronte degli unitari, perché l'idea unitaria, moderata, liberale e con Cavour non era l'idea democratica, repubblicana e centralista di Mazzini. Esisteva, inoltre, una questione istituzionale irrisolta, irrisolta, difficoltà all'interno dello stesso côté liberale: le ha ricordate il senatore Menardi, quando ha fatto presente che l'opzione di Cavour per una monarchia parlamentare era ben diversa dall'ortodossia di una monarchia costituzionale, che non avrebbe mai previsto una comunicazione tra Parlamento ed Esecutivo, che era stata di d'Azeglio, di Balbo e che certamente

geografiche di unire un territorio profondamente differenziato nei suoi ordinamenti, nonché nelle sue realtà economiche. Sotto questo aspetto va ricordato che la Destra storica, e coloro i quali lavoravano con Cavour,

e non per ideologia. Infine, ricordo la difficoltà maggiore, quella per la quale l'Italia è stato l'unico grande Stato moderno che si è costituito contro la Chiesa, contro la Chiesa di Pio IX, la cui apertura riformista era stata ripagata con l'assassinio del suo primo ministro, Pellegrino Rossi, e che Cavour,

credenti e non credenti e se proprio è necessario dare una definizione del suo atteggiamento - che in realtà non è possibile

Ebbene, queste sono state le difficoltà che Cavour è riuscito a gestire politicamente per arrivare al risultato dell'unità, partendo da un'idea di nazione, signor Presidente, che non è stata l'unica idea di nazione che ha albergato alle origini del nostro percorso unitario. L'idea di nazione di Cavour si fondava sulla centralità della persona aveva poco a che fare - lo dico con rispetto - con un'altra idea che invece si fondava sul binomio nazione-popolo: quella mazziniana. Non era un'idea idealista ma piuttosto un'idea empirico-costituzionale; non era un'idea intrisa di democrazia, ma piuttosto di libertà. E soprattutto, proprio perché aveva conosciuto le difficoltà della politica estera, l'idea di nazione di Cavour considerava l'unità come un punto d'arrivo da consolidare e rafforzare, spendendo il massimo delle energie nella politica interna, piuttosto che un punto di partenza

sconfitta e soccombente. Lo è stata certamente degli anni di fine secolo, quando, di fronte al nazionalismo imperante a livello europeo, in campo politico-istituzionale e, invece, all'esplodere del cosiddetto modello tedesco che si era affermato sulla punta delle baionette dopo Sedan, la competizione interna vide contrapposti, da una parte, i sostenitori di una nazione estrema che si faceva nazionalismo e, dall'altra, una forza nuova che aveva il suo principio di fondo non tanto nella nazione quanto nella classe; mi riferisco al nascente movimento socialista. All'interno di questa divaricazione e di questa radicalizzazione del conflitto, certamente a soccombere fu l'idea nazionale di cui Cavour, il suo liberalismo, si era fatto portatore. Certamente l'idea di Cavour soccombette ancora al momento dell'avventura in Libia e al momento della partecipazione alla Prima guerra mondiale (almeno a Caporetto). E soccombette anche nel momento in cui lo Stato liberale crollò a favore del fascismo. Perché, vede signor Presidente, dubito che il fascismo possa considerarsi un anti-Risorgimento, così come Salvatorelli ha pure autorevolmente sostenuto. Nel fascismo è stata presente l'idea di nazione risorgimentale, ma non certamente nella versione cavourriana. Così come, quando il fascismo cadde e si tornò alla democrazia, noi riacquistammo quella libertà che è componente essenziale dell'idea di nazione da cui Cavour era partito ma non riacquistammo l'idea di patria, a causa dell'8 dell'8 settembre e anche a causa del fatto che la libertà ci provenne soprattutto dagli alleati e, infine, a causa del fatto che i partiti prevalenti non avevano più le loro radici e il loro DNA nella stagione risorgimentale. signor Presidente, i limiti che a lungo ha dovuto subire l'idea di nazione, al punto tale che fu un siciliano il maggiore biografo di Cavour. Mi riferisco a Rosario Romeo, il quale, parlando del senso comune oltre che della storiografia corrente,

così poco produttivo e così infausto. Oggi abbiamo rivisto molte cose sia a livello di storiografia sia a livello di senso comune; non vorrei che cadessimo nell'errore contrario: pensare che l'Unità d'Italia sia stata una passeggiata senza comprendere il dramma, la fatica, la sofferenza che c'è stata dietro l'azione dei nostri Padri fondatori, innanzi tutto di Cavour e di di coloro i quali lo affiancarono: quella Destra storica grazie alla quale l'Italia si mise in cammino per una storia difficile ma che è ancora la nostra storia oggi. *(Applausi dai commemorare la figura di Cavour in un'epoca come la nostra, ancora troppo segnata dalle ideologie e da tensioni quotidiane tra i poli, è come respirare aria pura a pieni polmoni. Perché nella sua storia, umana e istituzionale, si misura la politica come strategia di lungo periodo, l'intesa declinata come fine ultimo e non come puro tatticismo, la pratica parlamentare come reale agire al servizio della nuova Italia, l'importanza per la classe dirigente di avere uno scopo da perseguire. Rievocare il primo Presidente del Consiglio porta a misurarsi con il carattere e l'azione di un conservatore, perché indubbiamente tale fu, dotato al contempo di un'autentica apertura mentale, frutto delle numerose esperienze vissute negli Stati esteri, e di una spiccata curiosità per i progressi economici, produttivi e sociali. Un conservatore sì, ma non un reazionario. Di più, un riformista che sapeva temperare con coraggio e passione i rischi derivanti dall'utopia e che invece cercò di prevenire le fisiologiche storture di un processo unitario come quello che riguardò l'Italia. Andando a sfogliare con la memoria i discorsi per Roma Capitale, pubblicati un anno fa e impreziositi dall'introduzione del compianto professor Scoppola, si resta colpiti dalla forza dei convincimenti di Cavour, dal suo profondo senso dello Stato, dalla qualità del suo agire pragmatico. «Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità la rafforzano, invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario la riducono all'impotenza». Ecco l'essenza del pensiero di Cavour in una delle sue frasi più celebri; ecco la sintesi che lascia esterrefatti per la sua straordinaria attualità. Con queste parole Cavour esalta quel giusto mezzo, vera stella polare della sua politica, del disegno strategico di un uomo, di uno statista, che non diventò mai ostaggio di tribuni o massimalisti della prima (e anche della seconda ora), né complice o utile idiota di un disegno reazionario *tout court*, portatore in sé di risvolti oscurantisti. Impossibile, sia da un punto di vista storiografico che politico, non menzionare i gravissimi attriti che Cavour ebbe con la Chiesa cattolica. Ma in questa sede preferiamo, e lo dico da cattolico, puntare la nostra attenzione sulla lungimiranza dimostrata al culmine della «crisi Calabiana» o sulla formula «libera Chiesa, in libero Stato» che racchiude una realistica visione del governo di una Nazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia nacque come Stato unitario di impronta liberale, grazie soprattutto alla guida di Cavour, una figura di politico e statista incentrata sulla realizzazione del progetto fin dai primi anni della sua brillante carriere politica. Sindaco ad appena 22 anni del Comune di Grinzane, carica che ricoprirà per quasi 16 anni, Cavour fece del processo unitario il suo fine ultimo. Abile tessitore di alleanze, venne più di una volta additato dai suoi critici come una figura di rara spregiudicatezza politica. Conscio della posta in gioco, Cavour rispondeva così ai suoi detrattori: «Non tengo, voi lo sapete, al potere per il potere. Tengo ad esso per fare il bene del mio Paese». Parole, c'è da ammetterlo, che nell'Italia di oggi non vengono pronunciate con la stessa frequenza. In Cavour era forte la convinzione, alimentata giorno dopo giorno, che le buone leggi migliorano il livello morale di un Paese; che lo sviluppo e la crescita politica di un intero sistema non possono essere disgiunti dai progressi economici e che per fare ciò bisogna inseguire necessariamente un progetto, avere un'ambizione superiore. Lo dimostrano i tre discorsi pronunciati davanti al Parlamento italiano a pochi giorni dalla sua costituzione, nella primavera del 1861. In discussione era la questione di Roma e dello Stato Pontificio. Cavour si trovava di fronte a un'alternativa apparentemente di impossibile soluzione: o attaccare il Papa, distruggendo l'alleanza con Napoleone III e probabilmente provocare una guerra con la Francia, o rinunciare a Roma Capitale. Cavour uscì dall'*impasse* alzando il livello del dibattito, ossia trasformandolo in una questione di superiore ordine civile e morale. Che Roma diventasse la capitale d'Italia era necessario non per motivi nazionalistici, ma perché era l'unico luogo simbolico che potesse accomunare e non dividere il Paese, un luogo di conciliazione. Ciò che noi quindi oggi celebriamo nel 150° della morte di Cavour è la sua figura di conciliazione, l'artefice della nostra unità, lo statista che seppe valorizzare il ruolo dello Statuto albertino ancorandovi il concetto di patriottismo, il valore della libertà con quello dell'indipendenza, la riforma politica con il benessere economico. «Era un genio, statista di carattere europeo ammirato persino da Bismarck, ma anche un uomo coltissimo che non ha mai smesso di studiare». Così uno storico, qualche anno fa, definì Cavour. una figura irripetibile, da sempre in fuga dal potere centrale che già 150 anni fa aveva tracciato la strada che l'Italia dovrebbe seguire, ancor di più in queste ore: «La grande politica - disse - è quella delle risoluzioni audaci». E la nostra Italia, lasciatemelo dire, oggi ne avrebbe un gran bisogno.

credo che per capire Camillo Benso conte di Cavour siano fondamentali alcuni dati biografici, così come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduta. Nasce in una famiglia patrizia torinese, ma non è il primogenito e, come cadetto, è costretto a inventarsi un'attività. Inizia allora la carriera militare come ufficiale del Genio, ma in gioventù, pur essendo stato allevato in un ambiente fortemente conservatore, entra in contatto con i liberali di Ginevra, città natale della madre. È proprio in quegli anni, con i primi soggiorni all'estero, che Cavour comprende l'abissale disparità politico-culturale esistente tra un Piemonte allora provinciale e sonnolento e le più progredite Nazioni europee. In breve tempo diventa un fervente ammiratore dell'Inghilterra. Pur essendo nobile di nascita, assorbe la mentalità operosa della nascente borghesia capitalistica e in economia diventa un convinto liberista. Intraprende una propria attività indipendente come imprenditore agricolo, cosa che gli consente poi di diventare Ministro dell'agricoltura e Ministro delle finanze nel Governo di Massimo D'Azeglio. Esaurita in tutta Europa la spinta rivoluzionaria del 1848, anziché indulgere nella pura e semplice difesa dell'ordine costituito e della struttura amministrativa e autoritaria di tante monarchie del vecchio continente, Cavour si trasforma in un entusiasta sostenitore del modello inglese, la monarchia costituzionale. Non era più il tempo di aggrapparsi al vecchio ordine, all'*Ancien régime*. Come liberale, ma anche come nobile che comprende il valore progressista della borghesia, Cavour sarà determinante nell'influenzare la stessa evoluzione politica della monarchia sabauda. Vittorio Emanuele II, a differenza dei Borbone e dei Lorena e superando una educazione reazionaria reazionaria tipica della corte sabauda, si trasformò, proprio grazie a Cavour, in "Re Galantuomo" assumendo con coraggio il ruolo di sovrano costituzionale e patriottico. E in questa evoluzione, politica e culturale di Vittorio Emanuele c'è tutta la grandezza di Cavour. Quando, poi, con le leggi Siccardi del 1850, come in altre monarchie costituzionali, si rese inevitabile lo scontro tra Stato e Chiesa, si determinò la prima vera occasione per l'esordio di Cavour in politica. È bene ricordare che le leggi Siccardi abolivano privilegi secolari del clero e venivano colpiti anche i patrimoni delle congregazioni ecclesiastiche. Le proteste e le e le manifestazioni di piazza dei vescovi erano state represse con fermezza al punto di arrestare l'arcivescovo Franzoni di Torino. Cavour, allora quarantenne, si era già fatto notare per le sue idee liberali e liberiste con alcuni articoli sul giornale "Il Rinnovamento". Entrato da poco alla Camera, si fece poi notare per la sua difesa delle leggi Siccardi, affermando contemporaneamente una duplice vocazione politica a tutela dell'ordine pubblico e a tutela della libertà e, quel che più conta, schierandosi nettamente a favore della laicità dello Stato. Fu facile, in quella occasione, era il novembre del 1852, realizzare quel "connubio", cioè l'accordo organico e funzionale tra destra, liberale e borghese, e sinistra, moderata e progressista. Oggi Cavour va ricordato per tanti motivi, per aver dedicato la sua vita a realizzare l'Unità d'Italia, ma Per le inevitabili analogie tra presente e passato, oggi non può essere sottaciuta la genialità e l'avvedutezza politica di una intesa, di un accordo, ovvero di un "connubio" tra oppositori che si realizza superando diffidenze, perplessità e scetticismi e che, però, approda alla però, approda alla finalità suprema del bene comune. Cavour ha governato il Piemonte per sette anni, durante i quali riuscì a trasformare lo Stato sabaudo in un Paese moderno capace di sostenere il confronto con i Paesi più progrediti d'Europa e capace anche di rappresentare un polo di riferimento sicuro per tutti i patrioti italiani che si battevano per l'unità della Nazione. Liberale e liberista in economia, stipulò trattati con l'Inghilterra, la Francia e con il Belgio, sviluppò la prima rete ferroviaria attraverso gli Appennini; creò una base militare nel porto di La Spezia. La sua vocazione cosmopolita si dispiegò in termini culturali verso due direzioni principali: quella filo-britannica, riconoscendo i meriti della monarchia costituzionale, e quella filo-francese collegando il Piemonte e la Savoia alla Francia. Quando, nel dicembre del 1852, Luigi Napoleone, con un plebiscito risuscita l'Impero e assume il nome di Napoleone III, è Cavour la guerra di Crimea che, con il successivo Congresso di Parigi del 1856 consentì al minuscolo Piemonte il diritto di sedere al tavolo delle trattative con le più grandi potenze europee e poi gli accordi di Plombières che precedettero la II Guerra d'indipendenza La strada per l'Unità d'Italia fu spianata dopo le più cruente battaglie del Risorgimento italiano, a San Martino della Battaglia, nel comune di Desenzano del Garda, e Solferino, del 24 giugno 1859; ma si doveva attendere ancora un paio d'anni prima della proclamazione dell'unità nazionale che stiamo celebrando nel 150° anniversario. Napoleone III lasciò Villafranca sottoscrivendo una resa che poteva essere spiegata, da un lato, con la volontà del monarca francese di consentire una espansione limitata del Piemonte e, dall'altro,

proclamazione del Regno d'Italia. Dal 17 marzo 1861 al 6 giugno successivo si svolse la residua parte della vita di Camillo Benso, conte di Cavour. Come evitare il rimpianto di una perdita così grande proprio quando l'Italia era appena nata? Qual è l'ammonimento che a 150 anni possiamo ricordare? Il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, lo abbia detto molto bene pochi giorni fa,

Cavour quando ha detto che la crescita di un'economia non scaturisce solo da fattori economici, ma dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse, dalla condivisione di valori e speranze. Gli stessi fattori determinano il progresso di un Paese. lei stesso ha ricordato il connubio tra risorgimento economico e Risorgimento politico. Al riguardo, scriveva ancora Cavour: «Il risorgimento politico di una nazione non va mai disgiunto dal suo risorgimento economico. Le virtù cittadine, le provvide leggi che tutelano del pari ogni diritto, i buoni ordinamenti politici, indispensabili al miglioramento delle condizioni morali di una nazione, sono pure le cause precipue dei suoi progressi economici». Occorre sconfiggere, quindi, gli intrecci di interessi corporativi che in più modi opprimono il Paese; è questa, in conclusione, una condizione essenziale per unire solidarietà e merito, equità e concorrenza, per assicurare una prospettiva di crescita al nostro Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi oggi vogliamo intervenire per commemorare il primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, Camillo Benso, conte di Cavour, di cui ieri è ricorso il centocinquantesimo della morte. Il capo della Destra moderata fu un grande riformista nell'amministrazione dello Stato italiano che andava a formarsi, fu promotore di idee liberali, del progresso civile ed economico con l'introduzione del libero scambio e il sostegno alla crescita della rete ferroviaria. Cavour fu un grande protagonista del Risorgimento italiano, quale innovatore culturale, un forte credente nel progresso soprattutto intellettuale e morale alla base della dignità dell'uomo. Il politico piemontese fu Ministro del Regno di Sardegna dal 1850 al 1852, Capo del governo dal 1852 al 1859 e dal 1860 al 1861. E' stato solo grazie al genio politico di Cavour, alla sua capacità di intessere alleanze antiaustriache, prima con la Francia poi con la Prussia, che dai rovesci militari si è arrivati alla riunificazione della penisola. Ma lo statista sabaudo ha avuto un unico difetto: morire troppo giovane, perché questa non era l'Italia che immaginava e sognava; il suo progetto era quello di creare un modello di Stato capace di unire e non semplicemente di unificare popolazioni divise da realtà storiche, politiche, culturali, produttive. Come ha più volte affermato il Ministro delle riforme per il federalismo, onorevole Umberto Bossi, «Cavour era federalista, la promessa e l'impronta federalista sono state fondamentali nel percorso dì unificazione del Paese. Senza questa premessa e senza questa impronta i Lombardi non ci sarebbero mai stati a finire sotto il Piemonte». Come hanno sostenuto altri studiosi: «Cavour era l'unico uomo politico dotato del carisma e dell'autorevolezza necessari per portare a termine la grande riforma federalista. Morto lui, la burocrazia e tutto l'apparato di potere del vecchio Regno sabaudo ebbero buon gioco nell'affossarlo». Secondo Cavour, il decentramento poteva unire meglio una penisola multietnica, come sostenne anche un altro padre del federalismo: Carlo Cattaneo. Così, il Primo ministro del Piemonte spinse il Ministro degli interni, Carlo Farini, a elaborare un disegno di decentramento. Il 24 giugno 1860 Farini istituì una speciale commissione in cui, per la prima volta, si parlò di Regioni e di Governatori. Scrisse Farini: «Stabiliti i limiti delle Regioni, dovranno essere determinate le attribuzioni. Ogni Regione è sede di un Governatore che rappresenta il potere esecutivo con le attribuzioni. Fanno capo a esso politicamente gli intendenti delle Province». A Farini successe poi Marco Minghetti come nuovo Ministro degli interni, che proseguì i lavori della commissione. Nella seduta del 28 novembre 1860, Minghetti inoltre sostenne che si potevano decentrare almeno quattro Ministeri: Interni, Istruzione, Lavori pubblici e Agricoltura. Il primo ministro Cavour, alla vigilia della proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861, conferì mandato al ministro degli interni Marco Minghetti di elaborare un progetto di riordino amministrativo ispirato ad un ampio decentramento. Su questa linea Minghetti elaborò un'articolata proposta, tendente a conciliare le esigenze del nuovo Stato con le esperienze e le tradizioni dei governi locali. Il Ministro ipotizzava sei grandi unità territoriali, le vere e proprie macro-Regioni. Queste aggregazioni avrebbero riunito, sulla base di un consorzio di carattere volontario e permanente, le Province affini per vicinanza territoriale, per storia, interessi, modelli culturali e tradizioni. Grazie alla dislocazione amministrativa, le Regioni avrebbero introdotto con gradualità e senza forzature gli ordinamenti dello Stato unitario, con l'obiettivo di armonizzarli con le antiche prerogative dei territori e delle comunità. Minghetti proponeva dunque un disegno realmente innovativo, del tutto inedito nel contesto europeo, per contrastare quella che Cavour aveva definito la «tirannia centralizzatrice». Il progetto Minghetti, presentato il 13 marzo del 1861, si scontrò però con l'opposizione frontale di una classe politica incapace di prendere in seria considerazione questa soluzione. Dopo un acceso dibattito parlamentare, l'esame del disegno di legge venne rinviato ad una commissione dove, contro di esso, si formò un largo schieramento di opposizione composto dagli esponenti della vecchia burocrazia piemontese, ma anche della sinistra fuoriuscita dai ranghi della fazione mazziniana che ne decretò la bocciatura, in ragione di una malintesa difesa del carattere unitario del nuovo Regno. Oggi il percorso federalista è ben avviato. Con 150 anni di ritardo piano piano la promessa e l'impronta federalista di Cavour si stanno realizzando. Come ha detto il nostro segretario federale, Umberto Bossi: «Oggi è arrivato il momento di riprendere quella promessa e mantenerla compiendo davvero la storia». Come disse lo stesso Cavour: «Per traversare una montagna che ci separa da una fertile pianura, bisogna fare lunghi giri per evitare i precipizi di cui il più sovente è seminato il cammino». La classe politica di oggi e di domani è a uomini e politici come Cavour che si deve rifare, a uomini che hanno saputo guardare al futuro con uno sguardo sognatore ma concreto; ed è a uomini con la sua stessa forza di volontà politica, ma soprattutto con la stessa forza morale, che deve ispirare le proprie azioni. signori senatori, voglio iniziare questa commemorazione ricordando che, senza l'opera e la personalità del piemontese Camillo Benso, conte di Cavour, forse l'Italia unita non ci sarebbe stata e per tutti noi sarebbe molto più difficile dirci italiani. Dobbiamo al genio politico di Cavour la straordinaria regia di quel complesso processo storico che nel 1861 portò a compimento l'unificazione della Nazione italiana. Nel poco tempo a disposizione non potrò fare né una completa biografia, né una agiografia di Cavour, né potrò eguagliare la mirabile commemorazione del professor Piero Craveri, ieri, alla Camera dei deputati. Per la biografia sarebbe difficile fare meglio di Italo De Feo e di Rosario Romeo, che di Cavour si sono tanto e così eccellentemente occupati: in particolare, Rosario Romeo, siciliano, come ha ricordato il senatore Quagliariello, e Cavour piemontese, a riprova dell'artificiosità di quanti oggi, per interesse politico, si ostinano a contrapporre gli italiani del Nord a quelli del Sud, non riuscendo a vedere quel che Cavour, 150 anni fa, aveva ben compreso, e cioè che a noi non servono due, tre o quattro Italie: a noi serve una Italia sola. Oggi il Senato è chiamato a ricordare e rendere onore a Cavour con parole non retoriche. Dobbiamo riflettere su cosa possa significare per noi la sua lezione politica e cercare di ricostruire un filo conduttore del suo pensiero, che ci consenta di approfittare delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e dell'anniversario della scomparsa di Cavour per valorizzare quanto di positivo c'è nell'Italia di oggi e correggere i nostri limiti. Insomma, l'anniversario di Cavour dovrebbe spingerci ad occuparci dell'Italia di oggi e di domani, delle sue divisioni, dei suoi giovani senza lavoro, del suo mancato sviluppo, della disuguaglianza profonda tra i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Se riusciamo a collegare Cavour al nostro presente e trarne una lezione per il nostro futuro, questo anniversario sarà stato utile all'Italia. Cavour comprese e governò la spinta all'unificazione, cominciata molto prima del 1861 e del Risorgimento, dando un naturale sbocco ad un lunghissimo processo culturale e sociale che doveva portare alla formazione della nostra identità nazionale. La Nazione italiana (non lo Stato, ma la Nazione), come comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dal senso di una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di Stati nei quali la penisola era andata via via variamente articolandosi, comincia a formarsi nell'età medievale. Si è chiusa da poco a Roma una piccola, ma straordinaria mostra, allestita al Palazzo del Quirinale, che di questo lungo processo ha dato un'impressionante testimonianza. Una mostra di manoscritti dei più grandi autori della letteratura italiana: da Dante Alighieri a Machiavelli, da Petrarca a Galileo Galilei, da Goldoni a Ugo Foscolo, da Alessandro Manzoni a Giacomo Leopardi. Al di là dell'emozione di vedere la scrittura di Manzoni sui «Promessi sposi» o di Leopardi su «L'infinito», la considerazione più importante che quella mostra ha suscitato nei visitatori è che quelle opere testimoniano che almeno dal 1200, da Dante Alighieri in poi, l'Italia era già unita nella lingua e nella letteratura. Dovremmo riflettere sul fatto che uno dei più consistenti ostacoli all'unificazione reale dell'Europa è tuttora la mancanza di una lingua comune. Ma, nonostante l'unità linguistica, fare l'unità d'Italia fu per Cavour un'opera ciclopica. Sette eserciti divennero un esercito solo. Furono tracciate le prime linee della rete ferroviaria nazionale. Furono organizzate le Poste nazionali. Fu creato un sistema severissimo di imposte per sostenere spese pubbliche crescenti e per pagare l'interesse del debito. che mi hanno preceduto, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Come fu possibile per Cavour portare a compimento in pochi anni quest'opera colossale? In primo luogo con la politica, e cioè con la suprema sapienza della sua guida politica, che rese possibile la convergenza verso un unico, concreto e decisivo traguardo di componenti politiche, sociali ed economiche molto diverse. Cavour comprese le necessità e le aspirazioni dei diversi Stati della Penisola, vide in seno a quelle società e nelle città italiane l'emergere di ricche e imprevedibili riserve, che seppero farsi eroismo nello slancio dei volontari. Erano sensibilità fatte di ideali, di cultura e di politica, risorse senza le quali nessuna grande impresa può essere possibile.

società in molte sue parti matura, classe dirigente all'altezza della sfida: proprio quel che oggi manca all'Italia! Ma il capolavoro di Cavour fu la sua comprensione del quadro internazionale e la sua capacità di approfittarne. Il processo unitario era "credibile" in Europa perché in Piemonte c'era Cavour. Lo dimostrano i risultati e i riconoscimenti che gli vennero in quegli anni dalla politica e dalla cultura europee; riconoscimenti del significato positivo che aveva per l'Europa la nascita di un'Italia unita e i riflessi che essa avrebbe avuto sulla storia di altri Paesi europei negli ultimi decenni dell'Ottocento. L'orizzonte europeo era al centro della visione e dell'azione politica di Cavour. Riflettiamo, signori senatori, su quanto grande e "concreta" possa essere per le Nazioni l'importanza del prestigio internazionale dei *leader* politici e su quanto pesi la coesione tra gli Stati. E pensiamo all'Italia d'oggi così in difficoltà nel credito internazionale! Un'altra mostra di straordinario interesse è tuttora in corso a Roma (molti di voi l'avranno visitata e a chi non l'ha fatto consiglio di andarvi) ben capire quanto poderosa fu l'intuizione unitaria di Cavour. È una mostra curata dalla Banca d'Italia che ha come oggetto «La moneta dell'Italia unita». motivo questa mostra ci deve interessare a proposito dell'opera unitaria di Cavour? Perché segna, anche quantitativamente oltre che qualitativamente, lo sforzo immenso di colui che ha costruito l'Italia unita. Nel 1861 le monete circolanti nei territori italiani unificati erano ben 236, alcune con corso legale, altre no; 282, se si considerano anche le province venete e romane che si unirono successivamente - come voi sapete - al nuovo Stato. Questa molteplicità di monete risentiva di fortissime stratificazioni storiche. Il processo di unificazione della moneta si concluse nel Centro-Nord nel 1865 e nel Mezzogiorno trent'anni dopo, per completarsi solo nel 1893-1894. Questo perché al Sud molte monete erano in argento e, poiché il prezzo dell'argento saliva, molti risparmiatori preferirono conservare le monete d'argento e cambiarle con la lira solo quando il prezzo cominciò a scendere. La riflessione sulle difficoltà incontrate nella nascita della lira deve far riflettere il Senato della Repubblica su come 150 anni fa l'Italia prima compì il processo di unificazione politica e solo dopo unificò la moneta. In Europa abbiamo fatto e stiamo facendo esattamente il contrario. Abbiamo l'euro ma non abbiamo l'unità politica. Forse non era possibile fare diversamente. Ma possiamo accontentarci di avere una moneta unica europea senza avere quell'unità politica che ne dovrebbe costituire la premessa? Concludendo voglio sottolineare come il ciclo governativo di Cavour abbia segnato l'inizio di un nuovo modo di governare, nel quale non c'era più posto per l'improvvisazione e l'inefficienza. Il valore di Cavour è stato riconosciuto anche dai suoi avversari politici più risoluti, e ne aveva tanti, a destra e a sinistra. è stato riconosciuto come un grande uomo di Stato, che in tutta la sua vita e in tutta la sua azione politica ebbe un unico obiettivo: quello di fare grande il suo Paese. Una concezione della Nazione non "popolo", come diceva il senatore Quagliariello, ma forse neanche una concezione di Nazione come "persona". Io penso che in Cavour esistesse una concezione di Nazione-Stato. Oggi, nel ricordare Camillo Benso, conte di Cavour, dovremmo prendere l'impegno solenne di far sì che l'interesse politico di parte di ciascuno di noi non prenda mai il sopravvento sugli interessi della Nazione. *(Applausi dal

È per la verità con particolare piacere che oggi invece rivolgo un saluto caloroso ad un giovane alpino di 99 anni, Antonio Porrini, di Besozzo, in provincia di Varese.

Per questa settimana rimane confermato l'esame del disegno di legge anticorruzione fino alla sua conclusione prevista per la giornata di giovedì 9 giugno. Peraltro, in relazione a richieste avanzate da alcuni Gruppi, con riferimento alla chiusura della campagna elettorale per i *referendum*, le votazioni termineranno alle ore 15. Nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 15, il Governo renderà un'informativa sui recenti attentati in Libano e Afghanistan che hanno coinvolto i militari italiani. Giovedì 9 giugno, alle ore 15, il ministro della salute Fazio renderà un'informativa sui rischi connessi alla diffusione del batterio *escherichia coli*. Sui due argomenti i Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno. Il calendario della prossima settimana prevede 1'esame dei disegni di legge sulla insequestrabilità delle opere d'arte e sull'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché della ratifica Italia-Marocco sulla cooperazione militare e delle mozioni Ramponi sulla sicurezza da minaccia cibernetica e Bertuzzi su una strategia mondiale per il settore alimentare. Mercoledì 15 giugno, alle ore 12, verranno poste in votazione le dimissioni reiterate dal senatore Nicola Rossi.

reiteratamente chiesta la fissazione dell'esame dei provvedimenti in materia di corruzione, presentati, per il mio Gruppo, nel giugno 2008 (penso analogamente per il Gruppo del PD),

hanno dovuto attendere, senza poter fare nulla, perché non veniva consentito di lavorare nel rispetto del Regolamento e quindi con i pareri Siamo arrivati quindi in Aula in una situazione del tutto singolare, anche se non rara: finalmente sono stati formulati i pareri sugli emendamenti, ma nel momento stesso in cui sono stati formulati, era era stata già fissata dalla Conferenza dei Capigruppo la discussione in Aula. Quindi, lo scorso giovedì noi abbiamo preso atto della realtà della fissazione in Aula e, in considerazione del gran numero di emendamenti formulati dal relatore,

peraltro tutti quanti d'accordo che il provvedimento andava implementato dalle iniziative emendative.

Gli emendamenti sono stati presentati sul disegno di legge del Governo. Si aggiunge poi un altro fatto:

il disegno di legge di ratifica, proposto dall'Italia dei Valori e dal Partito Democratico,

obbliga il nostro Governo ad adeguare la normativa interna a ciò che è contenuto nella Convenzione.

siamo arrivati in Aula senza relatore, oggi interviene un fatto nuovo.

Presidente, non intendo intervenire sulla funzionalità dei nostri lavori perché la questione che ci si pone oggi non è procedurale, né alcuno, ovviamente,

Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, che è ovviamente una ratifica che attende poi di essere tradotta in norme con le quali il nostro ordinamento si adegui a quelle

risposta a questa domanda il nostro lavoro, celere o non celere, funzionale o no, rischia di essere senza senso e credo che ciò sarebbe molto grave per un procedimento legislativo. Il problema è che emendamenti tendenti ad un adeguamento sulla base della ratifica della Convenzione di Strasburgo sono stati presentati sia in Commissione che in Aula. Sono emendamenti sui quali il Governo ha sempre espresso parere contrario, così come contrario è stato in Commissione il parere del relatore di maggioranza. sono contrari sulla base di un rapporto gerarchico o temporale, ma sulla base di una valutazione di merito: mi chiedo

poiché questo lavoro che riguarda la ratifica della Convenzione di Strasburgo si è già concluso positivamente in Commissione, non è forse ovvio che l'Assemblea, nell'affrontare il provvedimento sulla corruzione,

Si intende dunque che questo lavoro, cui noi attribuiamo una grandissima importanza, è un lavoro - come si dice con una brutta espressione - *in progress*, nel senso che approfitteremo del lavoro dell'Assemblea affinché ricadenti nel nostro ordinamento sulla base di quella ratifica, oppure no? Non è un fatto di metodo, non è un fatto procedurale, non è un espediente ostruzionistico. Dopo avere

cosa dice la maggioranza. Riteniamo di attribuire tutti a questo provvedimento la medesima importanza e quindi di farne «il» luogo, e non uno dei luoghi nei quali compiere a puntate quest'opera? Penso sia questa la domanda preliminare: non prendo neanche in considerazione lo dico subito - il ritorno in Commissione del provvedimento, perché come sempre è l'*animus* ad essere determinante. Abbiamo già assistito, nel corso di questa legislatura, al rinvio in Commissione di un provvedimento come la riforma la riforma dell'ordinamento forense, con il risultato che esso è rimasto un altro mese in Commissione e non è stata cambiata una virgola. Dunque, quello che conta è l'intenzione: abbiamo l'intenzione di fare tesoro di questo trovato di questo trovato consenso intorno a quella ratifica, oppure no?

La questione che ha posto la presidente Finocchiaro, che condivido, è di natura politica, prima ancora che procedurale. Su questo è evidente che la risposta non può darla lei,

Signor Presidente, onorevoli senatori, le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno dato inizio all'esame del disegno di legge del Governo n. 2156, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e dei disegni di legge congiunti nella seduta dell'11 maggio 2010. Il primo problema che si è presentato, subito dopo le relazioni introduttive dei senatori Malan e Balboni, è stato quello del coordinamento tra l'*iter* di queste iniziative legislative e quello dei disegni di legge nn. 850 e 2058, assegnati alle Commissioni giustizia ed affari esteri in materia di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione, problema che si è ritenuto di risolvere, anche sulla base delle indicazioni espresse dalla Presidenza del Senato, nel senso di limitare la portata dei testi all'esame delle Commissioni giustizia ed affari esteri esclusivamente alle norme di ratifica in senso stretto.

16 giugno 2010, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite hanno svolto un approfondito ciclo di audizioni informali, nel corso del quale sono stati ascoltati: le associazioni di categoria della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché l'Unione delle camere penali; il procuratore nazionale antimafia; magistrati con particolare competenza nel ramo, quali il procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco, il procuratore della Repubblica di Bologna, dottor Roberto Alfonso, il sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello dell'Aquila, dottor Davide Mancini, e il dottor Piercamillo Davigo, della Corte suprema di cassazione;

il capo dipartimento del servizio anticorruzione e trasparenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i presidenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; pubbliche; i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia, i rappresentanti della Confindustria, di Rete imprese Italia, dell'associazione nazionale costruttori edili e del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; il Presidente dell'istituto nazionale degli amministratori giudiziari e rappresentanti del comitato di coordinamento dell'alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero dell'interno e della Banca d'Italia, rappresentanti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Il 27 luglio dell'anno scorso è ripreso l'esame, ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti dapprima per il 27 settembre, e poi, su richiesta dell'opposizione, per il giorno successivo. In data 29 settembre 2010 è iniziata l'illustrazione degli emendamenti e, in considerazione dell'ampiezza di taluni e dell'ampia portata di alcuni emendamenti dei relatori, sempre su richiesta dell'opposizione, è stato fissato per il 6 ottobre il termine per la presentazione di subemendamenti. L'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti è poi proseguita nelle sedute del 6 e del 20 ottobre, nonché del 3 novembre 2010. L'esame è ripreso il 18 gennaio 2011, ma - anche in considerazione del fatto che la Commissione bilancio, che aveva espresso il proprio parere sul disegno di legge in data 4 novembre, non si era però ancora pronunciata sugli emendamenti - i relatori e il Governo hanno ritenuto in due occasioni di rinviare anch'essi l'espressione dei loro pareri. Finalmente, nelle sedute del 3, 29 e 24 maggio 2011 i relatori e i rappresentanti del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti e, contemporaneamente, è pervenuto il parere della Commissione Pertanto, le Commissioni riunite sono state convocate in data 1° giugno al fine di dare inizio alla votazione degli emendamenti. in considerazione della notizia che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per quella stessa mattina, si sarebbe pronunciata sulla iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei disegni di legge sulla corruzione già nella seduta di oggi, le Commissioni riunite, anche in considerazione dell'imminenza della Festa della Repubblica e del fatto che la campagna referendaria in atto avrebbe reso impraticabile una convocazione straordinaria delle Commissioni riunite nel fine settimana, hanno ritenuto di non procedere alla votazione dei numerosi emendamenti e quindi del mandato ai relatori. apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Berselli, non essendo stato concluso l'esame nelle Commissioni riunite 1a e 2a,

devo dire innanzi tutto che forse abbiamo pensato che la corruzione riguardasse solo l'Italia, invece è un problema che riguarda tutti gli Stati, sia quelli progrediti che quelli non progrediti.

iniziò Mani pulite. È estremamente preoccupante perché altera la concorrenza, che le imprese, anziché cercare di migliorare la propria organizzazione, la propria capacità, cercano il padrino o cercano di corrompere e, quindi, attraverso la corruzione superano tutti questi ostacoli.

funziona. Lo stesso funzionario che ha dato in concessione l'appalto, infatti, quando deve andare a controllare l'opera, se è stato corrotto e trova qualcosa che non va, non sarà certo lui a rilevarla. La corruzione finisce con l'incidere anche sulla qualità delle opere che vengono date in appalto. Detto questo, sottolineo che il problema della corruzione della corruzione affligge l'Italia in maniera particolare. Secondo una graduatoria di *Transparency international*, solo negli ultimi due anni, l'Italia è passata dal 55° al 73° posto, dopo il Cile, la Corea del Sud, il Costa Rica e addirittura il Botswana, che forse qualcuno non ha mai sentito nominare perché si tratta di uno Stato tra lo Zimbabwe e il Sudafrica con poco più di un milione e mezzo di abitanti. Allora, io mi domando: per quale ragione un Paese come l'Italia, che è certamente civile e che ha un'ottima polizia e un'ottima magistratura, si trova al 73° posto? Non so quanto sia attendibile questa graduatoria, però una cosa è certa:

La criminalità organizzata, infatti, disponendo di una quantità di denaro liquido immensa è in condizione di corrompere chiunque, non ha bisogno di minacciare.

Quale è la ragione fondamentale per cui la corruzione in Italia cresce? In questa Aula sono stato chiamato anche assassino per avere fatto Mani pulite. Me lo ricordo perfettamente, e mi è dispiaciuto molto, perché eravamo convinti che effettivamente si stesse facendo una cosa seria contro la corruzione. Infatti, badate bene, il potere politico, per ottenere che gli appalti andassero a finire a chi dovevano andare, ha dovuto servirsi della classe burocratica.

Ora, chi si è corrotto una volta, signora Presidente, si corrompe di nuovo. si corrompe di nuovo. È questo il guaio della corruzione, e perciò la corruzione in Italia è così diffusa. Ma allora, quale è la domanda che dobbiamo porci?

effettivamente combatte la corruzione? Effettivamente riduce la corruzione?

doveva cercare, innanzitutto, di uniformare le nostre norme giuridiche a quelle degli altri Stati che hanno sottoscritto le nostre stesse convenzioni, che ora sono state entrambe approvate: sia la Convenzione dell'ONU del 2001 sia la convenzione di Strasburgo del 2009, che abbiamo approvato oggi in Commissione all'unanimità. Cosa bisognava fare, innanzitutto? Creare un organo assolutamente indipendente per il controllo degli appalti, sia pubblici che privati, signora Presidente. Invece, cosa vogliamo fare con questo disegno di legge? Abbiamo creato un osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione,

Quindi, restano fuori dall'oggetto di questo osservatorio i contratti urgenti, che non seguono la normativa dei contratti pubblici. Restano fuori anche i contratti per le grandi opere, che non solo vengono sottratti al controllo preventivo della Corte dei conti, ma vengono anche sottratti a questo osservatorio. allora, se sia giusto che una legge che voglia effettivamente contrastare la corruzione affidi questo osservatorio, innanzitutto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli ultimi scandali ci dicono che, forse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva vicino persone, specialmente quando si parla di appalti di grandi opere, che forse non facevano tanto il loro dovere.

appena 40 giorni dopo che questo organo, assolutamente indipendente, finalmente aveva stipulato una convenzione con

non saranno inseriti né i contratti urgenti né quelli delle grandi opere. Ma istituire una banca dati,

per combattere la corruzione. D'altra parte, se si fare una cosa seria non si sarebbe neanche dovuto fare quello che è stato fatto per gli enti locali.

ma che dipendano dallo stesso ente il controllo sugli appalti che vengono stipulati e sui contratti pubblici credo sia una delle cose più inverosimili. È come se, per i contratti in cui si verifica la corruzione, non si rispettassero le regole:

il risparmio e dire: "Comunicate prima agli organi contabili che fate questo contratto, e se vi si dice che i fondi ci sono, lo fate", allora è tutto un altro discorso.

quando la pena è inferiore a sei anni, per calcolare la prescrizione si comincia dai sei anni. In sostanza, si è aumentata la pena, senza incidere minimamente sul termine di prescrizione. Non solo. Non si è modificato neanche l'articolo 158 del codice penale, che fu modificato nel 2005 proprio per evitare che, per calcolare la prescrizione in caso di corruzione, si partisse dalla fine della continuazione. e si continuerà in tal modo perché non è stato detto niente in questa legge - la prescrizione si calcola dalla consumazione di ciascun reato. ad immaginare un funzionario che si corrompe per 500 volte; la maggior parte dei reati, nel momento in cui viene scoperta, è già prescritta o si prescriverà durante il processo.

danni. Signora Presidente, quando un reato si prescrive, il giudice non può disporre la confisca neanche di quanto ha sequestrato. Quindi, se ha sequestrato ciò che ha ricevuto come compenso della corruzione, lo deve restituire.

con una crescita che nel 2010 ha registrato un aumento di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo *Transparency International*, nel decennio 2001-2010, con riferimento al parametro corruzione, l'Italia è scesa dal 29° posto che occupava, spostandosi dal gruppo dei Paesi democratici più avanzati e collocandosi in posizioni di coda nelle graduatorie internazionali, insieme a Georgia, Brasile, Guatemala ed Egitto. Le analisi internazionali relative all'impatto della corruzione sull'economia, assumendo come parametro di riferimento il *Corruption Perception Index*, ci dicono con evidente chiarezza che vi è un rapporto tra il prodotto nazionale lordo, il tasso di crescita del prodotto interno lordo, il costo del rischio di investimento, il costo del credito, il livello degli investimenti diretti esteri e il fenomeno corruttivo. Il costante sviluppo di questi raffronti evidenzia una significativa correlazione fra la corruzione ed i fattori indicatori della crescita economica del Paese. Proprio oggi, in un interessante convegno organizzato dalla Farmindustria di Sergio Dompè, si è offerta l'occasione per rilanciare nel dibattito pubblico il tema della legalità e dell'efficienza, termini sostanzialmente antinomici rispetto alla correlazione fra corruzione e spreco. La rilevanza e la drammatica attualità del tema è racchiusa in una recente dichiarazione del ministro Brunetta che rileva come il balzello occulto della corruzione «equivale ad una tassa di mille euro all'anno per ogni italiano, neonati

ha riflessi sulla cultura e i valori della società. Più del 70 per cento della società ritiene che nei prossimi anni la corruzione sia destinata a non diminuire. È di questi giorni il il rapporto del Consiglio d'Europa sulla corruzione in Italia, che si conclude con 22 raccomandazioni di valenza amministrativa che riguardano la necessità di introdurre standard etici procedurali per evitare l'interruzione dei processi e normative relative alle nuove figure di reato. Sulla base di tali sintetiche osservazioni non si può che salutare con particolare apprezzamento e convinta determinazione il disegno di legge oggi in discussione, le cui misure sono dirette a contrastare i fenomeni di corruzione sotto il profilo istituzionale, penale ed amministrativo, offrendo così un segnale chiaro e preciso al Paese e rispondendo ad una forte esigenza di trasparenza e di controllo sull'uso del denaro pubblico, confermata dallo stato di diffuso

e le buone pratiche di prevenzione della corruzione specificamente previste nel capo II della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU, con riferimento anche alle iniziative da intraprendere, che trovano riscontro nell'odierno provvedimento. provvedimento. Quest'ultimo rafforza l'efficacia dissuasiva delle norme penali ed agevola la repressione di fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale. Ma c'è di più: questo disegno di legge fonda la sua architettura anche su norme mirate alla prevenzione del fenomeno della corruzione e introduce criteri di selezione della classe politica, liberandola dalla mortificante condizione di casta e restituendole il suo significato più alto, come peraltro spesso in quest'Aula attraverso un lavoro faticoso e serio che svolgiamo insieme. La trasparenza dell'attività amministrativa, l'accesso e la conoscenza dei procedimenti da parte dei cittadini rappresentano fattori determinanti per favorire il controllo e la verifica della legalità dell'azione amministrativa. L'istituzione dell'Osservatorio sulla corruzione e sugli altri illeciti nella pubblica amministrazione e le numerose iniziative di medio e lungo periodo sono un ottimo viatico anche per adeguare l'ordinamento giuridico agli standard internazionali. L'approvazione di tali misure è indispensabile ed urgente, anche al fine di restituire al Paese e alle sue istituzioni quella necessaria credibilità a cui, purtroppo, i fenomeni corruttivi hanno inferto un duro colpo, con effetti negativi anche sugli investitori esteri, il conseguente rallentamento dello sviluppo economico, e l'estendersi La valenza del provvedimento è resa più evidente più evidente dalla crisi finanziaria, nella consapevolezza che i maggiori costi che derivano dai fenomeni corruttivi si riflettono direttamente sul debito pubblico e, in definitiva, sulla pressione fiscale cui sono sottoposti i cittadini. Trasparenza è, dunque, la parola d'ordine che deve aprire le porte al controllo ed alla responsabilità, con le sanzioni che sono lì a ricordare che «cosa pubblica» significa «cosa di tutti», come tale va gestita nell'interesse collettivo. Un monito, da questo punto di vista, arriva non solo dalla magistratura penale e da quella contabile, ma anche da altre autorità come quella sugli appalti pubblici, la cui attività di indagine conferma come, non di rado, l'esercizio dei pubblici poteri sia motivo di alterazione dei principi della concorrenza, con un possibile orientamento verso l'illecito utilizzo delle risorse pubbliche per coagulare in modo indebito il consenso politico o per ottenere indebiti benefici economici personali. Ma l'efficacia del disegno di legge in discussione appare di non meno rilevante efficacia anche per la semplificazione burocratica, perché uno snellimento delle procedure e una maggiore possibilità di interlocuzione dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione non possono che rivelarsi positivi sia ai fini della lotta all'illegalità e alla corruzione, sia della crescita e dello sviluppo. È proprio in questo senso questo senso l'istituzione presso le prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, con l'obbligo di un continuo aggiornamento delle liste, soprattutto per quanto concerne le società. Va osservato, infine, che i fenomeni corruttivi non sono solo quelli con evidente e conclamata valenza penale. Sì, perché esiste anche una forma di corruzione che talvolta si palesa si palesa in modo apparentemente privo di risvolti penali, ma che forse per questo è ancora più grave, perniciosa e subdola. Mi riferisco a quei comportamenti dei pubblici poteri che usano la burocrazia come strumento per l'indebito esercizio di un'azione discrezionale che è capace di complicare o di semplificare una procedura amministrativa, adattando i provvedimenti della pubblica amministrazione in funzione di appartenenze, di intrecci d'interesse e di inconfessate contiguità tra poteri di vario genere. Cosa dire poi, per esempio, dei piani di rientro? Questi sono disciplinati da norme ben precise stabilite in ambito nazionale, che poi in modo assolutamente abile, almeno in parte e troppo spesso, in periferia, a livello regionale, vengono disattese, per creare le condizioni che favoriscono evidentemente, in dispregio ad un patto sancito in ambito nazionale, condizioni per coagulare un consenso politico. Ecco perché non si può che apprezzare e condividere la norma contenuta nell'articolo 9, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del cosiddetto fallimento politico: si stabilisce, cioè, che i responsabili di sciatterie amministrative e gestionali, che determinano effetti dirompenti sulla corretta gestione delle risorse economiche, siano temporaneamente incandidabili per cariche elettive locali o nazionali e si dispone un ampliamento dei casi di scioglimento delle assemblee qualora non sia deliberato il dissesto finanziario. Una previsione che sostanzialmente conferma quanto stabilito dall'articolo 17 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo. Approvando questo testo noi non approviamo soltanto delle regole, a mio avviso facciamo molto di più: diamo al Paese un segnale importante con cui la politica, nei suoi livelli più alti di rappresentanza, conferma la volontà precisa di recuperare il principio della legalità come fattore irrinunciabile di crescita sociale ed economica, di rispetto per il merito e per i diritti individuali, di garanzia per gli stessi assetti democratici di un Paese che non può e non vuole evidentemente rassegnarsi alla cultura della corruzione, e dove essere onesti non porta - come talvolta accade - l'effetto avvilente di essere esclusi, ma di essere inclusi in un sistema virtuoso, che vuole partecipare della crescita comune del Paese. La legalità è un'opportunità. Speriamo, anzi siamo sicuri, diventi il punto di partenza per il riscatto delle nuove generazioni, senza dimenticare mai che davanti a noi possono esserci cose cose migliori di quelle che ci lasciamo alle spalle. Tocca anche a noi, tocca anche a quest'Aula volerlo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al pari di altri provvedimenti presentati dal Governo, anche questo, quando quando venne presentato nel maggio 2010, venne annoverato nell'ambito delle scelte cosiddette epocali. Ci siamo nutriti in questi anni di interventi epocali ed abbiamo nostalgia di qualche intervento legislativo normale al fine di evitarci il trauma di trovarci sempre dinanzi a delle svolte che cambiano la nostra esistenza. Senonché, il provvedimento presentato dal Governo è di una povertà assoluta, totale. La gran parte delle norme proposte riguardano alcuni ritocchi a norme già esistenti: si cambia qualche virgola, qualche nome. Poi vi è è tutto il capitolo che riguarda i bilanci dei Comuni ed il fallimento politico, ossia il dissesto finanziario, anch'esso introdotto già nel nostro ordinamento,

introduce le disposizioni per la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, fallimento politico, dissesto, e delle spolveratine sulle modifiche al codice penale, con minimi ritocchi di pena. Insomma, di fronte ad un fenomeno quantificato in 100 miliardi di euro, stimato per un costo per ciascun cittadino di 1.000 euro l'anno, noi rispondiamo con il niente. Rammento che intorno al problema della corruzione si sviluppano due correnti di pensiero; rimasi sorpreso diversi anni fa quando in un'aula di giustizia un alto ufficiale dei carabinieri

di quella che viene chiamata la trattativa all'indomani della strage di Capaci. E riferiva dei contenuti dei contatti con Vito Ciancimino. Ci riferiva il colonnello De Donno che, nell'ambito della trattativa, un capitolo riguardava la corruzione. Ossia, Vito Ciancimino, gli anni - riteneva che la nostra economia fosse destinata ad un rapido declino in quanto riteneva la corruzione funzionale alla crescita economica del Paese, facendo l'esempio - così come ci ha riferito il colonnello De Donno - di un'autovettura alla quale si sia tolta una delle quattro ruote. L'economia del nostro Paese non può cioè camminare senza corruzione. Tant'è che Ciancimino, vantando una grande onestà nell'ambito di una condotta disonestà e vantando altresì il fatto di essere stato sempre esente da critiche nel dispensare il prezzo della corruzione incassata, si propose come restauratore dell'Italia pre‑Tangentopoli e come collettore nazionale del prezzo della corruzione, offrendo in cambio allo Stato la possibilità di qualche operazione laddove il fenomeno avesse superato dei confini istituzionalizzati. Il giudizio del colonnello De Donno, espresso in un'aula di giustizia - che mi lasciò stupito - e reiterato in più occasioni,

C'è qualcuno nel nostro Paese che ha pensato, e che probabilmente pensa, che senza corruzione la nostra economia è destinata a soffrire. Ne consegue che un contrasto forte alla corruzione, considerata motore dell'economia, diventerebbe cagionevole per la salute economica del nostro Paese. Non vorrei che si fosse ispirato a questo filone culturale chi ha elaborato l'indecenza di questo disegno di legge. legge. Visto e considerato infatti che si tratta di una spolverata insignificante, significa che la corruzione è considerata qualcosa da istituzionalizzare, nei limiti fisiologici, e, quindi, non in quelle possibili deviazioni patologiche. Diversamente non sarebbe comprensibile come sia possibile - lo ricordava il collega D'Ambrosio - che si sia trattato in questo disegno di legge di ritoccare lievemente le pene, facendo in modo che tutte, nonostante i ritocchi, avessero un termine di prescrizione minimo, ossia sette anni e mezzo e, se poi va in porto la cosiddetta prescrizione breve, sette anni. Si tratta quindi di ritocchi insignificanti, nessuna apertura a ciò che noi abbiamo sottoscritto

Nessuna di quelle indicazioni è qui contenuta: dopo 12 anni siamo ancora arroccati a far finta di contrastare la corruzione, facendo un manifesto di titoli senza contenuti. Pertanto, così com'è, questo disegno di legge è una vergogna per il Governo e per i cittadini.

Purtroppo, dalla vostra parte c'è solo demagogia, ma il provvedimento in esame si rapporta e si confronta con tutti gli altri Paesi europei. Il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula contiene misure volte a contrastare la corruzione e l'illegalità nel settore pubblico. È la prima volta che un provvedimento così importante arriva in Aula

(mi rivolgo al senatore D'Ambrosio che è stato uno dei protagonisti dell'operazione svolta a Milano), che ha - di fatto - decretato la fine della cosiddetta prima Repubblica. Ma ancora oggi il fenomeno della corruzione sembra resistere al tempo e alle inchieste, ripresentandosi con le medesime dinamiche, sia pure con personaggi e circostanze diverse. La corruzione non appartiene ad un solo gruppo politico. È trasversale, colpisce i singoli cittadini, le associazioni, le attività lecite

della voragine delle finanze pubbliche e dell'allontanamento dei cittadini dalle istituzioni da cui non si sentono tutelati. È la «patologia massima», una degenerazione che produce vantaggi personali nell'esercizio di cariche pubbliche a svantaggio degli interessi della collettività. La corruzione nelle pubbliche amministrazioni resta un fenomeno molto diffuso in Italia. Le cronache di questi mesi e di questi giorni ne offrono innumerevoli esempi. Le statistiche internazionali ci pongono tra i Paesi europei a più alto tasso di corruzione. La corruzione amministrativa è l'aspetto più patologico della mala amministrazione, nella quale si comprendono tutti i casi di amministrazione non coerente con le finalità assegnate dalla legge. Il quadro normativo degli ultimi anni si è arricchito di numerose iniziative legislative, di cui alcune giunte a compimento ed altre ancora *in itinere*. La lotta alla corruzione, la trasparenza nell'attività amministrativa e il controllo sull'operato degli enti locali sono stati i principali obiettivi dell'attività governativa dell'attuale Governo di centrodestra che in passato ed oggi sta combattendo la criminalità anche in forma spicciola nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Da qui l'introduzione nel nostro ordinamento di strumenti di tutela giurisdizionale attivabili anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la previsione di uno stanziamento di 2 milioni di euro nella manovra anticrisi destinato proprio al funzionamento di quegli uffici che hanno il compito di sviluppare le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito perpetrate in tutti i settori della pubblica amministrazione e la conferma dell'assegnazione al Dipartimento della funzione pubblica del personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti già attribuiti all'Alto commissario anticorruzione. Ma è il disegno di legge anticorruzione che stiamo esaminando l'asse portante di una serie di disposizioni di grande novità e rilievo che vede al centro una pubblica amministrazione più efficace e trasparente. A completare il quadro rappresentato è intervenuta, in data 29 settembre 2010, l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 849 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la corruzione civile. Dopo un 2009 che ha visto rilevanti cambiamenti grazie alla ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione, nel 2010 si è vissuto, con insolita frequenza, il riproporsi del dibattito sull'effettiva indipendenza dell'Autorità nazionale anticorruzione. Nulla è immutabile e tutto è migliorabile, ma questo perpetuarsi, a volte accompagnato da tentativi ipocriti, non trasparenti, di modificare la situazione, appare non solo estremamente sterile, dopo che il Parlamento si è pronunciato con puntuale chiarezza pochi mesi prima, ma ancor di più dannoso, tenuto conto che non aiuta - sia a livello nazionale, sia sul piano internazionale - il processo di rafforzamento della credibilità di questo «punto di riferimento» che opera in Italia e che rappresenta il nostro Paese nella specifica materia presso le Nazioni Unite, l'OCSE e il Consiglio d'Europa. Il legislatore, con la legge n. 116 del 3 agosto 2009, ha designato quale Autorità nazionale anticorruzione il Dipartimento della funzione pubblica, al quale erano state trasferite in precedenza competenze e funzioni del soppresso Alto commissario, e ne ha statuito, sulla falsariga di quanto già accade nei più importanti Paesi occidentali, l'indipendenza e l'autonomia. Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo l'azione nazionale nella specifica materia, perché mentre assicura all'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione la forza, l'impegno, il peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, contestualmente prevede che, in concreto, dall'analisi dei risultati ottenuti, traspaia con immediatezza l'esclusiva finalizzazione dell'operatività all'attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale o economico, quali quelli lamentati in passato da diversi Alti commissari per la lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione. Molti degli altri importanti Paesi che hanno adottato una soluzione analoga, quali la Germania, il Belgio, l'Austria, la Francia, la Croazia, la Spagna e gli Stati Uniti, non presentano, come l'Italia, un sistema repressivo assolutamente indipendente, così come indicato nella nostra Carta costituzionale. Insomma, una differenza epocale rispetto al dettato della legge di ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione, che ne dispone direttamente, senza alcuna intermediazione di altri atti normativi, l'indipendenza e l'autonomia funzionale. Nella stessa strategia di intervento si collocano gli interventi approvati dal Consiglio dei ministri nel corso del 2010, tra i quali il disegno di legge n. 2156 al nostro esame. Il Capo I del provvedimento contiene misure per la prevenzione del fenomeno della corruzione, frutto di un cambiamento culturale, prima ancora che giuridico, e che riflette un approccio multidisciplinare, nel quale i tradizionali strumenti sanzionatori rappresentano solamente alcuni dei diversi fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa. Il Capo II contiene norme relative ai controlli negli enti locali. Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In questo quadro, gli articoli da 1 a 5 stabiliscono le iniziative, di medio e lungo periodo, che rispondono, da una parte, alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini, e, dall'altra, alla necessità di adeguare l'ordinamento giuridico agli *standard* internazionali, riducendo così il livello di corruzione nel nostro Paese. Del resto, la corruzione, nella sua misura effettiva e in quella percepita da imprese e cittadini, è un enorme danno alla credibilità del Paese, perché disincentiva gli investimenti, anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico. L'articolo 1 del disegno di legge istituisce il Piano nazionale anticorruzione. Si tratta di uno strumento che attua le politiche e le pratiche di prevenzione della corruzione specificatamente previste nel capo II della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116. L'adozione del Piano nazionale anticorruzione, come riportato nella relazione del presente disegno di legge, si rende necessaria anche a seguito della valutazione fatta, tra l'ottobre 2008 e il giugno 2009, dal Gruppo di Stati contro la corruzione organismo istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia fa parte dal 2007. Tra le altre raccomandazioni formulate, il GRECO ha invitato il nostro Paese ad adottare un Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e a riferirne dinanzi al Consiglio d'Europa il 31 gennaio 2011. Del resto, la maggior parte dei Paesi europei, come Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Irlanda e Polonia, hanno già implementato piani o strategie anticorruzione, sulla base della Convenzione ONU in materia. Il contesto internazionale, quindi, spinge perché sia adottata anche dall'Italia questa importante misura per la prevenzione e il contrasto della corruzione. La trasparenza dell'attività amministrativa, l'accesso e la conoscenza dei procedimenti da parte dei cittadini rappresentano fattori determinanti per favorire il controllo e la legalità dell'azione amministrativa. In questo quadro, come già previsto con riferimento ad altre attività della pubblica amministrazione, l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la trasparenza amministrativa rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. A tal fine, l'articolo 2 prevede l'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi «sensibili», quali quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera. Al di fuori di questi procedimenti, lo stesso articolo 2 prevede che le amministrazioni debbano, in ogni caso, realizzare il monitoraggio dei termini del procedimento amministrativo per individuare anomalie nell'azione amministrativa che possano costituire sintomi di cattiva amministrazione o di inefficienza amministrativa. L'articolo 3 introduce misure per favorire la trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici modificando l'articolo 7 del codice dei contratti pubblici. In particolare è prevista l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere *a)* e *d)*, e dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni, i programmi triennali dei lavori pubblici, l'elenco dei contratti pubblici affidati, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione di lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. La disciplina delle modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati nazionale è poi demandata al regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici. L'articolo 4 ha la finalità di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e, al tempo stesso, di garantire maggiore certezza pubblica all'azione amministrativa. In particolare, mediante modifica all'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, si introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare, cosicché le stazioni appaltanti possano procedere alla verifica del possesso dei suddetti requisiti direttamente presso la Banca dati, laddove la stessa contenga la relativa documentazione, senza richiedere la documentazione ai concorrenti. Inoltre, quale ulteriore misura di semplificazione e trasparenza, è inserito, all'articolo 74 del codice dei contratti pubblici, un nuovo comma che prevede che le stazioni appaltanti richiedano, di norma, l'utilizzo di moduli predisposti sulla base dei modelli standard, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Signor Presidente, concludo sottolineando l'importanza di questo provvedimento,

il Governo e il centrodestra hanno scritto quello che volevate voi del centrosinistra. È pertanto inutile fare ostruzionismo su un provvedimento che, secondo il centrodestra, è voluto non solo da quest'Aula ma soprattutto da tutti i cittadini italiani.

accompagnati dalla professoressa Esther Happacher, e studenti della Libera università di Bolzano, facoltà di economia, accompagnati dalla professoressa Stefania Baroncelli. A loro va il saluto e il benvenuto del Senato.

sentiamo sempre più parole che sconfinano; io le definisco ingenerose, ma bisognerebbe usare anche termini un po' più forti: non corrispondono alla realtà. Si sente in Commissione affermare una cosa, poi, in Aula, sentiamo l'esatto contrario. È vero che questo è un testo che forse è stato rallentato un po' nel suo *iter*

È vero, affrontiamo un tema che non è da poco, e proviamo almeno a frenare il grande problema dell'illegalità nel settore pubblico. I settori sono importanti: si parte inizialmente dai pilastri della prevenzione, Conosciamo amministrazioni che possiamo definire

Le amministrazioni, secondo noi, possono essere soltanto efficienti (e trasparenti, di conseguenza), oppure inefficienti e corrotte. Bene, facciamo di tutto per evitare che le nostre

Un'amministrazione non efficiente, un'amministrazione corrotta non c'è dubbio che produce effetti negativi a catena, tra i quali anche quelli di carattere economico: è disincentivante per uno Stato straniero investire in uno Stato che non dà garanzia; la stessa macchina e lo sviluppo interno sono rallentati dal fatto di non avere amministrazioni che rispondono in tempi certi e con risposte trasparenti e non alterate dall'illegalità. Sarebbe stato interessante rispondere direttamente al collega Li Gotti, perché stiamo rispondendo anche non a un obbligo, se vogliamo, internazionale, ma sicuramente ad un invito: la Convenzione delle Nazioni Unite ci invita a seguire delle buone pratiche per dare risposte al sistema amministrativo, ai cittadini, alle imprese, a chi si rivolge alle pubbliche amministrazioni. È proprio la Convenzione delle Nazioni Unite che noi indirettamente con questo testo rendiamo praticabile e trasformiamo in norme operative nel nostro ordinamento. Ricordiamo che già altri Stati lo hanno fatto: se questa è acqua fresca, dovremmo dire che Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Olanda, Polonia e così via, avendo adottato gli stessi nostri provvedimenti, hanno adottato acqua fresca e che non si è fatto sostanzialmente nulla. Credo non sia corretto fare tali affermazioni. Si introduce questo famoso Piano Piano nazionale anticorruzione: un piano bello, dettagliato ed articolato. Ogni pubblica amministrazione deve definire il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione nei propri uffici; deve trovare misure per fronteggiare il rischio che rileva; deve verificare delle procedure di selezione, formazione e rotazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (perché sappiamo come sia probabile creare aree di potere che poi si possono prestare all'illegalità)

Il controllo sociale avveniva su un sistema estremamente trasparente. Nell'opacità sappiamo che si nasconde tutto ciò che è illegale. Indubbio è che apparteniamo a società che stanno correndo, a società che non consentono più di fermarsi, approfondire e relazionarsi, al punto che rischiamo di non conoscere neanche chi abbiamo di fronte.

da comunitario a comunitario, il che faceva che tutte le cose rientrassero in un binario di legalità, perché questa oppressione da controllo impediva di comportarsi in modi illeciti. Qual è la parola d'ordine e magica? È trasparenza: dove c'è trasparenza, c'è controllo e dove c'è controllo ci sono meno forme di illegalità. È proprio nella trasparenza che che trovo il cardine di questo provvedimento. La trasparenza sull'attività amministrativa, attraverso l'accesso e la conoscenza di ogni provvedimento da parte dei cittadini, che rappresentano il fattore il fattore determinante per il controllo e la legalità. In questo modo il cittadino accede, ha la disponibilità di tutte le informazioni delle pubbliche amministrazioni e delle banche dati, interviene, formula domande e ottiene risposte anche in tempi estremamente rapidi.

che rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali addirittura garantiti dall'articolo 117 della Costituzione. Cosa viene introdotto per le pubbliche amministrazioni? L'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali tutte le informazioni relative a procedimenti amministrativi sensibili

non pubblica e non rende trasparente la sua attività si presume che ci sia già qualcosa che non funziona, c'è una presunzione di mala amministrazione. Fra i doveri della pubblica amministrazione vi è, per esempio, il rendere noto un proprio indirizzo di posta elettronica certificata dove il cittadino interloquisce, trasmette istanze

È prevista l'istituzione di una Banca dati dei contratti pubblici nazionali, che già a questo punto trova e dà un supporto all'attuale codice dei contratti pubblici, dove troveremo e ogni impresa potrà trovare i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, gli affidamenti, le imprese che hanno partecipato, i costi, gli scostamenti di costo tra il preventivo e il definitivo,

la storia di un affidamento, di una gara, di un appalto pubblico, in modo estremamente trasparente. Se qualcuno intravede qualcosa di anomalo lo segnala alla pubblica amministrazione, che sarà in grado di dare immediatamente le risposte. le risposte. Questo potrebbe sembrare un forte appesantimento per le procedure amministrative, ma non lo è, e lo dice la legge, perché non dovrà avere gravami né di costi né di personale, in quanto si utilizzeranno le risorse esistenti.

dove troveremo il possesso di tutti i requisiti delle imprese che parteciperanno, che produrrà alla fine il vantaggio per le imprese di non produrre sistematicamente gli stessi documenti, perché la verifica del possesso di questi la troveremo già

Troviamo interessante il fatto che si realizzi un sistema di controllo anche nei confronti dei subappalti, per evitare la parte esposta a a ciò che non era controllato ed era meno chiaro. Anche i subappaltatori rientreranno nelle normative antimafia e in tutto ciò che verrà espletato nei confronti della ditta principale

far poi funzionare le macchine della pubbliche amministrazioni. Mi riferisco al fallimento politico introdotto nel contesto delle operazioni legate alla riforma del federalismo fiscale.

L'incandidabilità è una cosa importantissima, perché risanare e trovare le formule per evitare i dissesti è

non prevede, fino adesso, nessuna conseguenza dalla mancata adozione da parte dell'organismo consiliare della relativa delibera, viene introdotta la se il consiglio comunale non sancisce il dissesto, perché omette di farlo o perché ha problematiche di pressioni interne, sarà il prefetto a poter intervenire

(si citano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, i servizi ispettivi della Guardia di finanza) e altri elementi che fonte certa. Pertanto, il prefetto, ravvisando queste situazioni di dissesto, sarà egli stesso ad avviare le necessarie verifiche. Mutano anche le condizioni per noi parlamentari, per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in merito alla ineleggibilità. Fino ad oggi, infatti, la sentenza

patteggiasse e il patteggiamento, non essendo considerato sentenza di condanna, consentiva di procedere tranquillamente in una carriera politica, qualunque essa fosse.

concerne due sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato riguardo ad un ricorso fatto da una SOA della Campania

sostanzialmente in libera concorrenza.

chi si aggiudica l'operazione finirà per non espletare nessun tipo di controllo perché non avrà nemmeno le possibilità di farlo in quanto

in costanza di una condanna definitiva; la terza attinente alla trasparenza dell'amministrazione pubblica e i controlli degli enti locali e, infine, la quarta, ossia la parte sanzionatoria che riguarda l'aumento e il ritocco delle cornici edittali di taluni delitti dei pubblici

Innanzitutto, per le misure di prevenzione al fenomeno della corruzione basta pensare che il Piano nazionale anticorruzione è rimesso all'attività di Governo.

Per quanto riguarda le misure di trasparenza dell'azione amministrativa, varie norme suscitano perplessità nel merito. Al di là dell'enunciazione di principio, si rinvia a provvedimenti successivi in molti casi vengono replicati principi già compresi nella legge sul procedimento amministrativo o nel codice dei contratti pubblici e non sono previsti stanziamenti finanziari, indispensabili per l'attuazione degli obblighi previsti *ex lege*. non concordo affatto con il senatore Divina perché, senza questi stanziamenti, nulla si può fare. Passo poi alle misure interdittive e alle incandidabilità. La normativa appare largamente insufficiente perché non cambia, se non in minima parte, il sistema vigente.

riforma del sistema penale, dove si elevano di circa un anno il minimo e il massimo edittale dei seguenti reati: peculato, in cui si innalza solo il minimo edittale; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione ai danni dello Stato; indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato; corruzione propria e impropria; corruzione in atti giudiziari; turbata libertà degli incanti; astensione dagli incanti; frode nelle pubbliche forniture.

edittale al peculato e alla corruzione in atti giudiziari - ma in linea generale le cornici edittali, così aumentate, non superano in alcun caso gli otto anni; si fa ciò, da una parte, per non attrarre detti reati nella seconda fascia del disegno di legge sul processo breve dall'altra parte, per aggravare, se possibile, il disastro prodotto dalla legge ex Cirielli del 2005 in materia di prescrizione e dalla quasi totale cancellazione del falso in bilancio, avvenuta sempre ad opera del Governo Berlusconi nella XIV

Vorrei ricordare che l'OCSE si è presentata pochi mesi fa al Senato della Repubblica, chiedendo di parlare con la 1a e la 2a Commissione, per avere spiegazioni del perché il Governo non voleva adeguare la legislazione. Sul punto al contesto europeo noi dell'opposizione abbiamo consegnato i nostri disegni di legge e abbiamo detto che nulla possiamo fare

ai richiami provenienti dall'Europa, dalle Nazioni Unite, dal Gruppo greco, dall'OCSE e dalle decisioni GAI. In particolare, non si tiene conto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia sottoscrivendo la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione nel settore penale

e non si rispetta l'Europa. In questo i Paesi del Terzo mondo sono particolarmente bravi: ratificano per primi tutte le convenzioni internazionali e poi se ne fanno beffa, esattamente come sta avvenendo in Italia Diversamente, i disegni di legge presentati dal Partito Democratico, tradotti in questa sede in emendamenti, sono rivolti a rendere più efficace l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione e, in generale, del malaffare nella pubblica amministrazione e nel settore privato,

soltanto rimarcare che di fronte all'atteggiamento del Governo, che aveva promesso di ratificare la Convenzione di Strasburgo e che è intervenuto con un piano straordinario che non ha nulla di epocale, siamo stati costretti a presentare vari disegni di legge, integrando sempre più

il Governo ha presentato una vera e propria strategia di guerra per abbattere la lotta alla corruzione. Ricordo il provvedimento sulle intercettazioni, la prescrizione breve, anche brevissima tutto ciò che è contenuto anche in altri disegni di legge apparentemente non affini: ad esempio, il disegno di legge n. 1440 che inibisce l'azione del pubblico ministero, oppure la riforma costituzionale che che sottrae costituzionalmente la polizia giudiziaria al pubblico ministero. Tutto ciò abbassa certamente il quadro e l'importanza della lotta alla corruzione, mentre il PD propone, oltre alle disposizioni che adeguano il nostro ordinamento

una diversa disciplina delle intercettazioni, una diversa disciplina degli appalti pubblici, legata in particolare ai grandi eventi ed alle ordinanze di Protezione civile ed ai controlli preventivi della Corte dei conti, il divieto di arbitrato, un'autorità indipendente per il controllo dei fenomeni corruttivi nel settore pubblico e privato in relazione alla Convenzione ONU, obblighi di trasparenza e codici etici, e una vera e propria previsione realmente ai partiti politici la responsabilità dei candidati che presentano, sia nelle elezioni amministrative che in quelle al Parlamento nazionale ed europeo.

che il Parlamento ed il Governo intervenissero di fronte a continue e ripetute occasioni di corruzione nel nostro Paese. Quest'ultima

privo di fattispecie reali e di pene severe, incompleto, in sostanza una resa alla corruzione. Avevamo un'occasione particolare, preziosa,

adeguandola alle capacità del nostro Paese di reagire, dimostrando agli italiani, alle imprese, ai nostri territori, all'Europa ed al mondo intero che l'Italia non è quel Paese che oggi è classificato agli ultimi posti per i livelli di legalità e che quindi è ai primi posti per indice di corruzione. Ci voleva un'altra risposta e non capirlo, attardarsi, fare melina, giocare d'astuzia, provare a confondere le carte con questo disegno di legge è il segno evidente di una crisi e di una decadenza, ma è anche il senso di una responsabilità che voi vi assumete, il Governo e la maggioranza si assumono. Il nostro Paese brancola nella penombra: molti approcci e pochi risultati. Vi sono diverse letture sullo stato dei malesseri che attanagliano l'economia e la società italiana; difficilmente troviamo analisi serie e rigorose, che mettano al centro la necessità della società italiana di dare un colpo d'ala alle sue lente dinamiche di crescita e anche di fiducia, per approcciare in modo diretto il rapporto tra legalità e sviluppo. Solo in questo rapporto il nostro Paese può diventare grande; solo nel rapporto tra legalità e sviluppo si può comprendere la devastazione che porta con sé la corruzione; solo così potremo capire quali risposte severe, rigorose, progettuali possiamo prevedere nel nostro ordinamento. Sono pari a 60 miliardi i costi della corruzione; 150 miliardi i fatturati delle mafie. Oggi è stato presentato da parte di Legambiente il rapporto sulle ecomafie, che ancora adesso si aggirano intorno a 20 miliardi di fatturato. In sostanza, bisogna capire che si può voltare pagina, che si deve voltare pagina, che è necessario fare in modo che sulla corruzione ci sia la stessa tensione, lo stesso approccio che abbiamo avuto prima nei confronti della lotta al terrorismo, (come una vera minaccia per la nostra democrazia, come una pietra d'inciampo per la crescita del nostro Paese) e poi, seppur più lentamente, seppur con molte contraddizioni, nell'approccio alla lotta alla mafia. Anzi, considero la corruzione l'altra faccia della presenza mafiosa, e spesso i due fenomeni si mescolano, spesso l'uno nutre l'altro, spesso insieme costituiscono una forza dirompente che si abbatte sulle nostre economie, sui cittadini, sui territori, sulle stesse istituzioni locali. Avete previsto nel capo I tre momenti: un Piano nazionale anticorruzione, la Rete nazionale anticorruzione, l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione; tutti e tre in capo all'Esecutivo, tutti e tre sotto il controllo del Governo. Questo è Italietta! Cari rappresentanti della maggioranza, caro rappresentante del Governo, nei Paesi avanzati, quelli a democrazia matura, non si danno queste responsabilità direttamente in capo ai Governi. I Governi devono applicare buone pratiche di anticorruzione, devono avere la capacità di prevenire e di colpire, ma chi controlla, chi stabilisce cosa bisogna fare e come bisogna farlo e che soprattutto verifica i risultati, nelle democrazie avanzate è un organo terzo, al di fuori dei controlli della pubblica amministrazione. su questa vostra impostazione il nostro no è netto, il nostro no è deciso, e questa vostra impostazione fa crollare tutta l'impalcatura - tra l'altro molto debole, fragile - che avete costruito. Inoltre, rappresentanti della maggioranza e del Governo, sugli appalti potevate fare solo una cosa buona che da tempo vi si chiede, che la Commissione antimafia in diverse relazioni e con diverse maggioranze ha proposto al Parlamento, ossia la riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Come si può avere un controllo di legalità quando nel nostro Paese ci sono circa 30.000 stazioni appaltanti? La corruzione vince a priori, la corruzione si fa sistema, la corruzione si abbatte sulle opere pubbliche e sui cantieri e impedisce al nostro Paese di decollare su questo nevralgico aspetto dello sviluppo della vita sociale ed economica.

ed una per Regione per le grandi opere, potrebbe essere una risposta moderna ed efficiente. Ci sono oggi i numeri, le professionalità amministrative e le capacità per avviare un buon controllo sulle stazioni appaltanti, così come sulle gare al massimo del ribasso: stanno distruggendo l'economia, il sistema d'impresa, la capacità realizzativa che hanno sempre caratterizzato la cultura industriale delle nostre imprese di costruzioni e stanno mettendo in ginocchio le imprese sane, quelle pulite, quelli che rispettano le regole, quelle che denunciano le organizzazioni mafiose. Anche su questo non c'è nessun riferimento; anche su questo fate finta di non sentire e di non vedere e vi rendete responsabili di un vero e proprio disastro. Infine, Presidente, ci sono alcune questioni che riguardano alcuni punti molto importanti, che cito solo perché sia il senatore D'Ambrosio sia la senatrice Della Monica le hanno poste. Mi riferisco alla cosiddetta incandidabilità. Il codice etico della Commissione antimafia ha creato un osservatorio, che denuncia una continua lesione. Ecco perché bisognava approfittare di questo provvedimento per inserire quelle norme severe di incandidabilità che sono contenute nel codice etico della Commissione parlamentare antimafia e che non riguardano solo i reati contro le mafie, ma anche i reati contro la pubblica amministrazione. Lo stesso si può dire sulla durata delle pene; con quella durata delle pene e senza prevedere quelle fattispecie che qui sono state indicate - cito per tutti l'autoriciclaggio ed il falso in bilancio - non possiamo assolutamente avere un sistema improntato a severità. Negli altri Paesi la corruzione è la violazione etica del fondamento costitutivo dello stare insieme e così dovrebbe essere anche nel nostro Paese, visto che abbiamo un'ottima Carta costituzionale e siamo a 150 anni dall'Unità d'Italia per cui dovremmo finalmente rinnovare profondamente la nostra condizione sociale ed economica. Ecco perché il nostro no è serio e rigoroso. È un giudizio forte e motivato. E quindi faremo valere le nostre ragioni in Parlamento e nel Paese. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo ed i colleghi rimasti in Aula.

«Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di capire la differenza». Troppo spesso in politica ci barrichiamo dietro quella serenità e quella accettazione, dimenticando il coraggio che oggi è più che mai necessario per riuscire a ricostituire onestà e trasparenza, proprio a partire dall'amministrazione pubblica, nella *res publica*, per liberarla da quel malcostume e quindi orientarsi la sua aulica accezione etimologica. La trasparenza e l'onestà, infatti, sono le premesse necessarie ed imprescindibili per poter essere politici o amministratori, ma soprattutto per garantire ai cittadini

il giudice Piercamillo Davigo, che oggi è consigliere della Corte di cassazione. In un suo libro egli scrive che gli "strappi alla legalità sono di per sé un disvalore e devono quindi essere perseguiti e processati".

Un disvalore che colpisce non solo l'economia del Paese, ma che è capace di minare anche il processo democratico, trasformandosi in una misura premiale per chi non rispetta le regole. I fenomeni di concussione e corruzione, infatti, sono ormai diventati una patologia del nostro Paese perché non sono più l'eccezione.

che nel 2010 i reati corruttivi sono aumentati del 30,22 per cento! Viene la pelle d'oca a leggere questi dati e sorrido perché mi sembra che il provvedimento che stiamo discutendo oggi sia inadeguato per affrontare questa emergenza. Il procuratore generale della Corte dei conti, Mario Ristuccia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2011 ha infatti lanciato un allarme, dichiarando che questi dati non consentono ottimismi e che la corruzione continua ad affliggere la pubblica amministrazione. Nel dettaglio della relazione della Corte dei conti si legge che nel 2010 sono stati denunciati 237 casi di corruzione, 137 di concussione e 1090 di abuso d'ufficio. In più, se noi guardiamo come siamo percepiti all'estero, il *Corruption perception index,* annualmente a partire dal 1996 dall'organizzazione non governativa *Transparency international* che ordina i Paesi del mondo sulla base del livello secondo il quale l'esistenza della corruzione è percepita

ci stia osservando e dica: «Ma per l'ennesima volta, oggi il Parlamento è incapace di leggere e di affrontare i problemi che si trova di fronte?».

Le cause di questo allarmante fenomeno sono profonde e non possono prescindere anche da un'interpretazione squisitamente antropologica del fenomeno e, quindi, dalla sfiducia nelle istituzioni, che comporta il non rispetto delle stesse a scapito della collettività e del bene comune. Se è vero che occorre intervenire per arginare questo fenomeno, non si può non considerare la larga fascia di cittadini onesti (e sono la maggioranza) che subiscono, loro malgrado, le conseguenze della minoranza. Infatti, i circa 40 milioni di contribuenti versano *pro capite* circa 1.500 euro di tassa occulta aggiuntiva, aggiuntiva, una somma che non dovrebbero versare nelle casse dello Stato e che invece sono costretti a versare a causa della corruzione e della concussione.

e sui loro capitali le imposte e le tasse. È un circolo vizioso, per cui la sfiducia verso le istituzioni comporta fenomeni di malcostume che, a loro volta, generano nuova disaffezione nei cittadini. Di fronte a questo triste scenario emerge che le norme esistenti nel nostro ordinamento non risultano in grado di spezzare questa catena e di favorire *in primis* un cambio di mentalità, che faccia della trasparenza l'unica soluzione possibile per trasformare quel circolo statico in una staffetta virtuosa. Gli stessi operatori del diritto e la giurisprudenza da tempo ammettono la necessità di una radicale riforma da questo punto di vista. Al riguardo, io stessa ho presentato un disegno di legge che forse

"I doveri dell'Uomo": "poco importa che voi possiate dirvi puri: quando anche poteste, isolandovi, rimanere tali, se avete a due passi la corruzione e non cercate combatterla, tradite i vostri doveri». Noi ce l'abbiamo a due passi da noi, anzi magari anche qui, allora dobbiamo sfruttare meglio questa opportunità e modificare questo disegno di legge.

e siccome non sono un addetto ai lavori del settore giustizia non posso mettermi a gareggiare per competenza con loro che, peraltro, hanno già spiegato benissimo perché questo disegno di legge è completamente insufficiente rispetto al fenomeno corruttivo.

era costretto a registrare, dalla lettura del dispositivo del provvedimento, che chi l'aveva scritto non aveva idea di cosa fosse la corruzione. spiegato in breve che mancava la percezione della connessione strettissima che c'è tra corruzione e concussione. Da lì si è poi dilungato a spiegare la corruzione come reato seriale, che avvinghia a sé anche gli inconsapevoli e alla fine costruisce una rete, il cui controllo risulta veramente molto difficile.

una legge anticorruzione prodotta da una maggioranza e da un Governo guidati da una persona che ha, purtroppo per lui e purtroppo per noi, una frequentazione ossessiva di procedimenti che riguardano reati di natura corruttiva. Lui se li vorrebbe scuotere di dosso; io, di fronte alle tante falsità che sono state dette su questo passato ingombrante e un po' offensivo per la natura stessa della Repubblica, ne traggo soltanto qualche scampolo, perché non potrei farne l'elenco completo. Ricordo un processo per la corruzione

Gli avvocati della Fininvest Previti, Pacifico e Acampora sono stati condannati per aver corrotto il giudice Metta, che ha annullato il lodo Mondadori, a vantaggio del proprietario precedente.

Di fronte a questa relazione così stringente tra il Presidente del Consiglio e i reati di natura corruttiva, ci si può stupire che la legge prodotta dalla sua maggioranza e dal suo Governo risulti così labile nel toccare tutta la rete dei fenomeni corruttivi? Non ci si può stupire. si può stupire. È stato ricordato che il lavoro della Commissione è stato vano e che per mesi ha lavorato a vuoto: in Commissione sono state rigettate tutte le proposte dell'opposizione, tutti gli emendamenti, tutte le soluzioni più incisive sul fenomeno corruttivo. Ricordo alcuni temi, ad esempio la relazione strettissima tra concussione e corruzione: Davigo ci spiegò che spesso il concusso è altrettanto corrotto del corruttore, anzi, ne trae un utile specifico e lo rinnova; il traffico di influenze illecite, la questione dell'autoriciclaggio e quella dell'incompatibilità tra ruoli di governo e

Non si tratta di una condanna definitiva, ma i colleghi dell'Aula potranno porsi il problema se il collega Grillo ha ancora titolo per mantenere la Presidenza dell'8a Commissione? Non sarebbe il caso che che si defilasse rispetto a certi ruoli? Il collega Divina ci invita a fare paragoni con la Germania. Ricordo che per il solo sospetto di aver utilizzato in modo improprio finanziamenti pubblici per la campagna elettorale, il *leader* della riunificazione della Germania, il cancelliere Kohl, è stato fatto fuori non dalla magistratura ma dal suo partito, che ha ritenuto che una figura come la sua, anche soltanto toccata da uno scandalo di cui non c'era nemmeno la prova provata in processo, non potesse più restare al proprio posto. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che fa collezione di procedimenti per reati di natura corruttiva e siamo nell'immobilità più assoluta. Non ci si può stupire di questo esito, perché mentre sui temi di interesse governativo, (vedi le leggi *ad personam*) il Parlamento viaggia a velocità supersonica, per leggi come queste ci impiega un anno per non fare praticamente niente: il Governo non fornisce pareri che avrebbe dovuto fornire alla Commissione, la 2a Commissione viene investita a raffica di nuovi procedimenti che ne inceppano il cammino.

che gestisce le grandi opere in maniera del tutto opaca, generando reti di affari, di speculazione, di corruzione e concussione e, di fronte a questo, siamo

una pallida sembianza di quella che dovrebbe essere una vera legge anticorruzione, per cui di fronte a questo prodotto il nostro giudizio non può che essere il più fermo e negativo possibile.

la catastrofe dell'inizio degli anni '90 sembrava aver posto fine alla questione morale.

rispetto al passato, forse perché la politica non se ne è voluta o potuta occupare a sufficienza. Recenti fatti di cronaca testimoniano come il fenomeno della corruzione è ancora nella vita politica e amministrativa del nostro Paese che affrontare il tema con qualche operazione di *maquillage*, di immagine, nascondendo la polvere sotto il tappeto, non farebbe certo bene al Paese. È pleonastico - lo hanno fatto meglio di quanto possa farlo io i colleghi che mi hanno preceduto - sottolineare come i fenomeni di corruzione siano fonti di inefficienza sul piano economico, di distorsione della concorrenza e come incidano nello sviluppo produttivo, e questo tenda a favorire indirettamente anche lo sviluppo della criminalità organizzata. Ci chiediamo allora perché un disegno di legge presentato in Consiglio dei ministri il 1° marzo 2010, sulla spinta elettorale delle amministrative e il dilagare degli scandali, annunciato poi il 4 marzo 2010 in Parlamento e esaminato nelle competenti Commissioni per oltre un anno, arrivi in Aula solo ora, sollecitato, vorrei ricordarlo al collega Cardiello, da tutta l'opposizione al completo. Voglio tranquilizzare il collega Cardiello: l'opposizione non vuole mettere bastoni tra le ruote a questa normativa, perché l'abbiamo sollecitata noi per un anno intero.

E come essere d'accordo con il senatore Divina - che io rispetto - quando parla di una buona legge e di qualche ritardo? Il senatore Divina dimentica, se non altro, che l'aspetto finanziario non è stato proprio toccato in questo disegno di legge. Il Parlamento è messo nelle condizioni di esaminare la questione con un gigantesco, colpevole, ritardo, che tutti abbiamo denunciato; eppure, nel frattempo, le grida di allarme non sono mancate: penso al richiamo del procuratore generale della Corte dei conti all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011; a proposito di corruzione e di frodi e soprattutto in materia di aiuti e contributi nazionali e dell'Unione europea egli ha usato questa definizione: «patologie che continuano ad affliggere la pubblica amministrazione». I dati non lasciano spazio all'ottimismo, come ricordato dalla collega Baio: nel 2010 la corruzione è aumentata del 30,22 per cento. Ma il dato più allarmante, se vogliamo, è il calo delle denuncie, quasi ci si fosse abituati al fenomeno, arresi ad una vera e propria cultura della corruzione; è come se la nostra società non sapesse più reagire con riprovazione morale ma dimostrasse uno spirito di rassegnazione, talvolta persino di accondiscendenza. Le maggiori preoccupazioni si concentrano nel mondo della sanità, ove malaffari e cattiva gestione imperano, aggravati da una carenza del sistema di controllo. L'importo complessivo del danno erariale contestato ammonta a 250 milioni di euro, in gran parte concentrato nella Regione Lazio (130 milioni di euro) e questo per frodi nella gestione di case di cura convenzionate e per irregolari erogazioni di prestazioni riabilitative. Se questa è la situazione e se questa maggioranza dichiara di volerla risolutamente affrontare, allora viene spontaneo chiedersi come si concilino la determinazione e il rigore necessari nella lotta alla corruzione con una serie di provvedimenti legislativi assunto in fase di gestazione da parte di questo Esecutivo. Lo stesso procuratore generale della Corte dei conti ha espresso viva preoccupazione per una serie di recenti interventi legislativi, tra gli altri il disegno di legge sulle intercettazioni (che costituiscono uno dei più importanti strumenti investigativi utilizzabili contro i fenomeni di corruzione) o la cosiddetta legge Cirielli del 2005. Le difficoltà nel perseguire i reati di corruzione sono state aggravate dalla riduzione dei termini di prescrizione e lo sarebbero ancora dalle forme anticipate di estinzione previste nel disegno di legge sul cosiddetto processo breve, di cui si discute in Commissione. La magistratura contabile ha inoltre espresso perplessità anche nei confronti del progetto federalista. Ci si interroga - cito testualmente - in termini dubitativi se il decentramento della spesa pubblica possa contribuire a ridurre la corruzione, ovvero possa avere l'effetto contrario e aumentare la corruzione quando la vicinanza a interessi e *lobby* locali favorisca uno scambio di favori illeciti in danno alla comunità amministrata. Pensiamo poi al frequente utilizzo da parte di questa maggioranza di procedure in deroga alle regole ordinarie, alla parificazione dei grandi eventi alle emergenze, che sottraggono i relativi appalti, bilanci, controlli al vaglio preventivo della Corte dei conti. Che dire poi del falso in bilancio? Purtroppo dal 16 aprile 2002 è operativa la riforma degli illeciti penali amministrativi delle società commerciali, di cui al decreto legislativo n. 61 Non aiuta certo a combattere la battaglia contro la corruzione, poi, la soppressione dell'ufficio dell'Alto commissario

Le informazioni rese al riguardo dal Governo sulle ragioni di tale decisione appaiono contraddette dal fatto che il servizio anticorruzione e trasparenza, oggi presso il dipartimento della funzione pubblica, risulta ancora privo di dotazioni adeguate dal punto di vista delle risorse umane e strumentali. un organo cui manca, inoltre, la necessaria autonomia per svolgere la propria funzione e che, in base alle relazioni presentate al Parlamento, mostra anche una preoccupante carenza di meccanismi propri di acquisizione conoscitiva. A ciò si aggiunga il ritardo del nostro Paese nella ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, che solo oggi è stata approvata, sia pure con modifiche. Siamo di fronte all'ennesimo piano nazionale che, in linea generale, ci appare carente ai fini del contrasto alla corruzione e richiede, al contrario, misure coerenti, risposte serie e concrete. Per questa ragione ritengo quanto mai opportuno istituire un organo indipendente che coordini l'attività di indagine e di contrasto del fenomeno, riservandomi di presentare a tal fine un organico disegno di legge. Tale organo di coordinamento risulta oggi necessario in quanto, nonostante gli sforzi dell'ordine e della magistratura, molti corrotti e corruttori riescono ancora a farla franca e pochi sono gli atti corruttivi portati alla luce, al punto che l'Italia è al 63° posto subito dopo la Turchia e a pari merito con l'Arabia Saudita, una posizione tale da spingere il Consiglio d'Europa nell'ottobre 2009 a dichiarare «molto seria» la situazione italiana. Siamo al 67° posto nel mondo. Tanto per capire, fanno meglio di noi Stati come il Cile, Israele, Turchia, Tunisia e Ruanda. Lo stesso Presidente della Corte dei conti ha evidenziato che «la lotta alla corruzione deve fondarsi essenzialmente su quattro pilastri: l'etica, la trasparenza, la semplificazione e il controllo». Per questo abbiamo presentato una nostra proposta legislativa. A monte di tutto ciò, però, occorre rispondere a un'esigenza di regolamentazione dell'accesso alla vita pubblica: la permeabilità di tale snodo procedurale ai meno nobili intenti è una delle peggiori ricadute della fragilità dell'attuale sistema dei partiti. L'attuale disciplina penale e processuale dei reati contro la pubblica amministrazione appare, infatti, inadeguata rispetto all'atteggiarsi concreto del fenomeno sotto vari punti di vista: anzitutto, l'apparato sanzionatorio risulta banalmente blando rispetto all'impatto sociale ed economico di reati di tale tipo, atteso che i responsabili in più occasioni hanno pagato con periodi limitatissimi di detenzione e, spesso, rientrando nel circuito della pubblica amministrazione in breve tempo; in secondo luogo, appare necessario aggiornare il catalogo dei reati utili, inserendo nuove ipotesi quali quelle di traffico di influenze di influenze e di corruzione nel settore privato, recependo così le indicazioni della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, che impegnava gli Stati aderenti all'esecuzione. Con tali norme si estenderebbe la punibilità penale di fatti di millantato credito e si introdurrebbe la nuova ipotesi della corruzione del privato funzionario, fino ad oggi solo teorizzata ma di fatto priva di una specifica copertura penalistica.

Inoltre, i rapporti illeciti tra criminalità e amministrazione pubblica possono facilmente svilupparsi con ingressi "secondari" di soggetti pericolosi nell'apparato amministrativo pubblico, tramite collaborazioni e consulenze di ogni genere; d'altro canto, il sistema corruttivo ha più volte prosperato attraverso la cooptazione dei controllori (si pensi a tutte le magistrature) con lo strumento degli incarichi extragiudiziari che, talora molto ben retribuiti, possono rappresentare il mezzo per legare controllori a controllati e per serrare un sistema di rapporti. Ci auguriamo, dunque, che l'esame in Aula sia proficuo, che non si sia chiusi, da parte di questa maggioranza, alle numerose proposte fatte dall'opposizione e che, insieme, si possa arrivare a correggere un testo assolutamente perfettibile e ad approvare il disegno di

il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione è stato sicuramente per il passato, ma lo è ancora oggi, un grosso problema nella vita sociale del nostro Paese. La proposta iniziale del disegno di legge puntava a modificare le previsioni del codice penale e inaspriva le relative pene. Il testo che oggi ci apprestiamo ad approvare risulta invece integrato in maniera diversa, con una serie di norme, elaborate dai ministri Calderoli e Maroni, che mirano invece a prevenire i fenomeni corruttivi in maniera forte e decisa, al contrario di alcuni interventi che ho ascoltato dall'opposizione. Il Governo ha voluto approvare un'ampia normativa, non solo sull'aspetto sanzionatorio ma anche a favore dell'efficienza della pubblica amministrazione, sanzionando il pubblico amministratore, a volte poco fedele, utilizzando come strumenti per combattere la corruzione, la semplificazione, l'efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione, introducendo il semplice ma efficace principio del chi fa cosa e, soprattutto, con la certezza di come e quando queste cose si fanno, l'identificazione certa del soggetto operatore, la certezza della procedura e della tempistica di ottenimento delle risposte, rendendo maggiormente lineari i processi decisionali nell'ottica della trasparenza amministrativa, chiaramente nell'interesse dei cittadini. Questo disegno di legge ha tre capisaldi: il Piano nazionale anticorruzione e trasparenza per ridurre i rischi della corruzione nella pubblica amministrazione; la disciplina degli enti locali, in cui vengono rafforzati i controlli e dettati i criteri di eleggibilità nelle cariche elettive; la definizione di norme sanzionatorie. Il Piano nazionale anticorruzione è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base dei singoli piani di azione predisposti dalle amministrazioni centrali, nei quali dovrà essere chiaramente indicato *in primis*, il grado di esposizione al rischio di corruzione dei propri uffici; le misure organizzative necessarie a fronteggiare tale rischio; le procedure di selezione; la formazione e rotazione dei funzionari che operano in settori sensibili; da ultimo, le soluzioni, anche normative, per prevenire ed individuare tempestivamente gli illeciti. È poi prevista una rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, che dovrà definire e fornire al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l'idoneità degli strumenti adottati, per definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici al fine di favorire il corretto esercizio delle funzioni ad essi affidate e monitorare costantemente l'effettiva attuazione dei singoli piani di azione. Ciò presuppone un ampio lavoro che la pubblica amministrazione dovrà fare al suo interno, al fine di dotarsi di segnali di allarme e di sensori (qualora le cose non funzionino adeguatamente) e di strumenti valutativi sui suoi dipendenti, forse per la prima volta responsabilizzando il pubblico amministratore in maniera da conferirgli il ruolo e la centralità che gli competono. Con questo Con questo provvedimento si realizzerà presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e di informazione. Le pubbliche amministrazioni dovranno concorrere con il principio della trasparenza, ovvero dovranno pubblicare sui siti istituzionali tutte le informazioni relative a procedimenti amministrativi "sensibili" (quelli cioè che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera). Le stazioni appaltanti dovranno trasmettere, tempestivamente e direttamente all'Autorità di vigilanza, tutti i dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di realizzarne la relativa anagrafe,

Un altro argomento molto importante è quello del controllo sugli enti locali, che avverrà migliorando i controlli sugli stessi enti sia sul piano della funzionalità, che della spesa.

è previsto che nei casi di rimozione del Presidente della giunta regionale, disposta ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, chi abbia ricoperto la carica di Presidente della Regione non possa essere candidato ad alcuna carica elettiva, né ricoprire incarichi di Governo o di amministrazione in enti pubblici nazionali o locali. E' ampliato l'insieme delle sentenze definitive di condanna che sono ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e relativamente alla assunzione di importanti cariche negli enti locali. Sono poi aggravate le sanzioni penali previste per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Stiamo parlando di una vera rivoluzione sul piano dei principi che dovrebbero ispirare i criteri del buon governo della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione finalmente aperta al cittadino, che trova gli anticorpi al suo interno per espellere quei funzionari che non si comportano in maniera molto deontologica. Ciò comporta una riflessione profonda e un mutamento di filosofia che ribalta il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino per introdurre finalmente la cultura del «servizio civile». Dirigere la pubblica amministrazione, o meglio dirigere nella pubblica amministrazione, significa affrontare con competitività un tema da sempre al centro delle riflessioni, del dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione in Italia, una pubblica amministrazione che con l'utilizzo delle nuove tecnologie riesce a dialogare con le aziende e le imprese attraverso la banca dati dei lavori pubblici e ad essere - speriamo - più competitiva e più moderna, finalmente in linea con gli altri Paesi europei. L'anima del disegno di legge si muove su un piano di prevenzione, di organizzazione e di analisi, che considera come ipotesi marginale la repressione, immaginando che le contromisure che la pubblica amministrazione adotterà serviranno a prevenire il fenomeno corruttivo piuttosto che a reprimerlo. Meglio, quindi, prevenire che curare. Non va poi dimenticato che il presente provvedimento è un mezzo attraverso il quale vengono attuate le politiche previste dal Capo II della Convenzione dell'ONU, adottata dall'Assemblea generale nell' ottobre del 2003 e firmata nel dicembre del medesimo anno anche dall'Italia.

detto altri colleghi, dal GRECO (gruppo di Stati contro la corruzione), anche in considerazione del fatto che già in molti Paesi europei sono state adottate queste misure anticorruzione. disegno di legge è in perfetta sintonia con la filosofia di questo Governo che da sempre ha lavorato in tale direzione, ricercando criteri di eccellenza nelle competenze sia dei dirigenti che dei funzionari che operano quotidianamente nel settore pubblico, anche attraverso la riforma della SSPA (Scuola superiore della pubblica amministrazione). La corruzione è in Italia un fenomeno che spaventa, soprattutto per il gran numero di piccoli episodi, diffusi in maniera capillare, che dilagano nella pubblica amministrazione e che causano un pesante danno erariale, oltre ad incidere sull'affidabilità che il cittadino inevitabilmente riconduce allo Stato come titolare della cosa comune. I fenomeni di corruzione minano sicuramente la credibilità dell'apparato pubblico e lo rendono perciò maggiormente penetrabile anche alle influenze criminali di tipo associativo. I fenomeni corruttivi vanno perseguiti con rigore, perché incidono sicuramente con conseguenze profondamente negative sulle amministrazioni,

Questo fenomeno porta ad una disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Occorre perciò muoversi su un piano etico e culturale, iniziando a lavorare all'interno dei dipartimenti dello Stato, consapevoli che la corruzione si annida maggiormente dove non c'è trasparenza

Occorre quindi rispettare le regole, essere chiari con i cittadini, osservare i tempi dei contratti e la regolarità delle contabilizzazioni nella gestione degli appalti, per evitare un ingente spreco di risorse pubbliche. Trasparenza e rispetto della legge sono chiaramente le condizioni per un uso corretto delle risorse pubbliche. Come abbiamo prima sentito affermare dal senatore Serra che mi ha preceduto, il nostro Paese non e' messo molto bene in quella classifica stilata

Tutta l'azione di Governo è quindi caratterizzata da scelte etiche riferite ai pubblici amministratori. In proposito voglio ricordare il codice di autoregolamentazione proposto nella relazione al Parlamento dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia,

18 febbraio 2010, un documento nel quale ha voluto impegnare tutti i partiti dell'intero arco parlamentare dall'astenersi nel presentare come propri candidati quelli in odore di criminalità, coinvolgendo anche i Presidenti delle Regioni, i sindaci e i Presidenti delle Province che a loro volta dovranno impegnarsi per effettuare le nomine in maniera uniforme ai dettami cui facevamo prima riferimento.

deve rendere attori e protagonisti tutti gli uomini che dirigono l'apparato statale, per realizzare una gestione della cosa pubblica finalmente senza sprechi ed inefficienze, ma produttiva e competitiva in linea con gli *standard* europei di cui

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta per le consuete "comunicazioni di servizio", ma in questo caso

che si sono recati agli sportelli dei servizi postali per richiedere le più diverse ma per loro essenziali operazioni, come riscuotere la pensione, pagare bollette di imminente scadenza piuttosto che la retta mensile dell'affitto, talvolta per alcuni anche in regime di sfratto esecutivo, considerato che un eventuale ritardo di pagamento, se non in grado di determinare l'imminente esecuzione per morosità, è comunque fonte di forte apprensione. Ebbene, lo spettacolo in cui sono stati involontariamente coinvolti i cittadini non è stato certo degno di un Paese che vorrebbe fare della modernità e dell'innovazione tecnologica la cifra della riforma per la trasformazione della pubblica amministrazione. Fuor di metafore e paradossi, si è verificato che un ordinario aggiornamento dei sistemi di *software* ha determinato un blocco dei servizi, che perdura tuttora, senza che siano state fornite adeguate spiegazioni ai cittadini sui motivi delle cause che hanno generato disservizi né tanto meno sui tempi in cui tali disservizi si sarebbero risolti. Al di là del fatto che non si comprende come una struttura così complessa come Poste Italiane, che fa del proprio sistema informatico ed operativo il proprio punto di forza, non disponga di un sistema di rete alternativo da poter attivare in caso di emergenza, come la circostanza attuale, sorprende la singolare coincidenza delle operazioni di aggiornamento con il pagamento delle pensioni che, per la maggioranza dei pensionati italiani, costituisce l'unica e scarsa provvista per il sostentamento della propria miseria condizione. Sorprende ancor più che, rispetto ai disservizi che si sono determinati, Poste italiane si sia distinta ancora una volta per improvvisazione, approssimazione e talvolta anche scortesia da parte del personale allo sportello, non posto nelle condizioni adeguate a fronteggiare disagi di simili proporzioni: 14.000 sportelli coinvolti, file chilometriche, con tempi di attesa di ore, spesso infruttuose e ripetute per giorni, in locali spesso privi di sedute o di servizi igienici, senza climatizzatori o non funzionanti. Dopo i dispacci di questi giorni diffusi da Poste italiane, in cui si fornivano sommarie ed inadeguate spiegazioni sull'accaduto e si dava per imminente la soluzione del problema, oggi sono finalmente giunte le scuse agli italiani dell'amministratore delegato di Poste italiane, ingegner Sarmi, per i disagi con l'annuncio che l'azienda si farà carico dei danni provocati. Ebbene, signor Presidente, apprezziamo il gesto, ma non basta, perché sull'accaduto vogliamo avere parole definitive di certezza. Ad oggi, la soluzione del problema è ancora lontana dall'essere intravista, come ci riferiscono continuamente e direttamente i disarmati operatori di sportello. Prevediamo purtroppo che ancora domani sarà una giornata di particolare travaglio. Non basta soprattutto perché occorrono parole di verità sull'accaduto, che siano in grado di diradare le molte ombre che si addensano sui processi di finanziarizzazione delle grandi imprese italiane - e Poste italiane lo è a buon titolo - che, in ragione di tali obiettivi, finiscono per smarrire vistosamente la propria missione sociale e la propria ragione industriale. Peraltro, se Poste italiane deve costituire, secondo le intenzioni del Ministro dell'economia con la propria rete informatica la struttura portante per la Banca del Sud, non è certo sotto i migliori auspici che si apre questo processo così importante e delicato. Ed è proprio per queste ultime, ma - comprenderà, Presidente - non secondarie ragioni, che chiediamo alla Presidenza del Senato di farsi interprete di tali richieste e di far disporre nella Commissione di merito, come peraltro abbiamo già richiesto al

finestra"). Senatore Filippi, la denuncia del disservizio che lei ha fatto ci ha visto tutti o coinvolti direttamente o interessati, potendosi

Noi abbiamo varie proposte di modifica del nostro Regolamento ma, da una ricerca fatta, risulta che l'articolo 148 non è interpellato per essere rivisto da nessun senatore presente. senatore presente. Sottolineo all'attenzione della Presidenza - forse non vi sarà sfuggito - che sabato scorso il quotidiano «La Stampa» ha pubblicato una durissima requisitoria contro i lavori della Camera e del Senato, conteggiando i minuti, le ore e i giorni di lavoro. Spero che la Presidenza, o chi per essa, abbia voluto interloquire con questo stesso articolo. Se però applicassimo il nostro Regolamento, questo lavoro di sindacato ispettivo, che non affronta quisquilie localistiche ma talvolta questioni di assoluta rilevanza, potrebbe impegnare meglio i nostri lavori e soddisfare meglio le esigenze di rappresentanza delle massime istituzioni a cui la

dovremmo tutti quanti riuscire a dare la versione giusta e comunque una risposta giusta.

finanze e delle politiche europee), riguardante il calcio scommesse. In questa interrogazione, signor Presidente, ho elencato una serie di partite che oggi sono oggetto di inchieste, partite segnalate e descritte, individuando anche i flussi anomali

apre una nuova finestra"). Anche questo è un tema di grande attualità, che in questi giorni sta colpendo molto l'opinione pubblica ed anche gli appassionati di sport che vorrebbero